Presidente, desidero comunicare all'Aula che ho da poco presentato un testo 2 dell'emendamento 91.850 (che insiste, appunto, sull'articolo 91), quale reca, oltre ad alcuni aggiustamenti di dettaglio, una diversa disciplina del regime transitorio riguardante il limite alle retribuzioni dei dipendenti pubblici. un regime transitorio che riprende alcuni subemendamenti presentati nella serata di ieri: in particolare, si prevede la non operatività della norma sui contratti aventi natura privatistica in corso e si disciplinano con un regime transitorio le altre tipologie di contratto e le altre retribuzioni, anche derivanti da cumulo di incarichi, attraverso una decurtazione graduale della quota eccedente il limite fissato del 25 per Ho altresì depositato un testo coordinato che rende più agevole la lettura. Ricomponendo l'emendamento con il testo originario, esso rende più agevole la lettura della complessa norma a cui mi sto riferendo.

Per poter giudicare, però, se si tratti di una riformulazione ovvero di un nuovo testo, e quindi se vi sia la necessità di apporvi eventuali ulteriori subemendamenti, attendiamo che il testo ci venga distribuito.

Presidente, mi associo a quanto detto dal presidente Schifani, sottolineando anche il profilo regolamentare della procedura alla quale stiamo assistendo. quale stiamo assistendo. Ieri abbiamo assistito ad un singolare duetto tra il Ministro della giustizia e un importante ed autorevole Presidente di Gruppo della maggioranza

dice la maggioranza, al di là del testo che qui viene presentato, e capire su che cosa verte la ricomposizione. Credo inoltre che in presenza di un nuovo emendamento - perché così lo ha presentato il relatore - ci sia un dovere d'illustrazione seria per capire che cosa prevede la normativa. Se ho ben capito, si rinvia, così come si dice in dialetto «a babbo morto», l'applicazione della stessa.

Presidente, i colleghi intervenuti mi hanno anticipato. Anch'io chiedo una sospensione dei lavori per valutare questo emendamento che stiamo leggendo in questo momento, mentre mentre stiamo parlando. Quindi, chiedo una sospensione congrua per poterlo esaminare. Presidente, io non mi limito a chiedere la sospensione congrua. Pongo in evidenza una situazione paradossale: noi, Gruppo UDC, abbiamo presentato ieri, sulla base di quanto era stato detto,

Si metta d'accordo una volta per tutte! Ci dica qual è il testo finale, veramente finale, e noi presenteremo gli emendamenti. Altrimenti continuiamo a fare bagatelle. Ieri il collega Antonio Boccia ha parlato dell'opposizione in termini offensivi. Noi come opposizione vorremmo sapere con chi abbiamo a che fare, collega Boccia! vorremmo sapere con chi abbiamo a che fare, collega Boccia! Per esempio, si parla dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili: che significa che un magistrato non può avere più del presidente della Corte di cassazione? Lo dico anche alla collega Finocchiaro, che è un magistrato. Il riferimento ai magistrati Il riferimento ai magistrati è ai magistrati che conosciamo, o è altra cosa? Noi non possiamo andare avanti così, Presidente, lo dico per la dignità del Senato. Il termine deve essere serio, ma pretendo - pretendo! che il relatore ci dica qual è la posizione finale della maggioranza. Signor Presidente, naturalmente condivido quanto ha detto il senatore D'Onofrio e non credo che basti, senza un chiarimento, una congrua sospensione. Peraltro, questo è un tema che è nel comune sentire della gente, è nella sensibilità della pubblica opinione; non so bene con quale

in modo plebiscitario, insieme con - quella sì - una casta che vorrebbe prendere il posto del Parlamento (e per un parlamentare, scusatemi tanto, associarsi a questa è veramente una vergogna), e poi non accettare l'emendamento Polledri,

non chiede soltanto una sospensione, ma intende approfondirne le motivazioni. Chiedo soprattutto a lei, Presidente, di far uscir fuori in via definitiva dalla maggioranza una posizione in relazione alle vicende che riguardano la parte economica di chi gestisce la cosa pubblica, perché sono in totale difformità.

La situazione mi sembra abbastanza chiara e piuttosto semplice anche da risolvere. Siamo in presenza di un emendamento del relatore al testo dell'articolo 91 della legge finanziaria. Come io stesso ieri ho avuto modo di dire nel corso della seduta che ricordiamo, si trattava, e si tratterebbe anche adesso, di dare un tempo, congruo a mio giudizio, perché i Gruppi possano esaminare il nuovo testo proposto dal relatore, relatore, con quelle motivazioni che egli qui ha portato, in modo da consentire l'eventuale presentazione, da parte di ciascun Gruppo, se lo ritiene opportuno, dei relativi subemendamenti. Questa è la situazione; non è che stiamo discutendo adesso, senatore Cutrufo, del merito dell'articolo 91, questo lo faremo dopo. Vorrei dire però ai Vorrei dire però ai Capigruppo delle forze politiche di opposizione che sono intervenuti che, a proposito della coesione politica o meno, a proposito del grado di convincimento o meno o meno della maggioranza, e ovviamente del Governo, sul testo dell'articolo 91 e sull'emendamento che è stato presentato dal relatore, c'è solo un modo Anziché stare qui a continuare a parlare di questioni metodologiche che a questo punto, se mi permettete, non hanno né capo né coda, procediamo ad una sospensione della seduta, dando tempo ai Gruppi di presentare subemendamenti

linea di massima (naturalmente poi si vedrà: la maggioranza è molto composita, complessa e giustamente articolata e dialettica al suo interno) comunque rappresenta il parere del relatore, della Commissione bilancio, dell'intera maggioranza e del Governo. Quindi, presidente D'Onofrio, è questo il testo sul quale anche le opposizioni dovranno confrontarsi, votare ed eventualmente dimostrare se la maggioranza è veramente unita o no. Personalmente rivolgo al presidente Storace) che sia una norma di grande importanza. Presidente Cutrufo, io non ho mai parlato di casta, mai; lo fa chi in genere va in televisione e ha una cattiva idea della politica e in genere anche un doppio linguaggio, nel senso che parla di casta in televisione e poi difende in quest'Aula tutti

l'opposizione: ho fatto rilevare soltanto che c'era un impegno a dimezzare gli emendamenti e che ciò non è avvenuto; non mi pare un'offesa. Per il resto, signor Presidente, come hanno detto gli altri

La seduta è ripresa.

Presidente, in tutto l'*iter* di questa finanziaria abbiamo sempre assunto un comportamento di grande responsabilità e, contrariamente a quanto accaduto l'anno precedente in occasione della manovra

abbiamo presentato per l'Aula un pacchetto minimo di proposte emendative, il più basso della storia parlamentare;

contro quelli che dovrebbero essere gli atteggiamenti di confronto con i parlamentari da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento - aveva indicato il numero di emendamenti

Non abbiamo accettato questa proposta, ma abbiamo ulteriormente ridotto le nostre proposte emendative. Abbiamo lavorato in Aula senza fare ostruzionismo; ci sono stati confronti decisi e articolati

vi è un intero testo di legge, non un articolo, quindi, che mette in discussione alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento e della nostra esperienza giuridica. È lungi da noi l'idea di non affrontare il tema della riduzione dei compensi dei pubblici amministratori, eliminando alcune storture,

Vengono avanzate proposte che cambiano ogni giorno, perché purtroppo, signor Presidente, la maggioranza,

a quella che prevedrebbe che i contratti di assicurazione in essere, stipulati regolarmente nella logica della piena autonomia negoziale di una società di assicurazioni,

la convocazione immediata di una Conferenza dei Capigruppo, perché su questo testo occorre una nuova articolazione dei lavori d'Aula, dal momento che è un nuovo testo di legge che merita un grande approfondimento. Se così non fosse, naturalmente non ci staremo e saremo costretti, signor Presidente, a venir meno, non per nostra responsabilità,

c'è una vicenda incredibile, perché il testo che ci è stato presentato stamattina non è un emendamento e nemmeno un articolo di legge. Ha ragione il presidente Schifani: qui siamo di fronte a una nuova legge

non può avere *cachet* pagati da nessun'altra parte dello Stato. Caro Russo Spena, ti voglio fare questo esempio: un insegnante di un conservatorio guadagna 1.300 euro al mese.

che si possa andare avanti: chiedo che si sospendano i lavori e che si riunisca una Conferenza dei Capigruppo perché prima di tutto dobbiamo rimodulare i tempi, dal momento che vogliamo approfondire questo articolo e discutere gli emendamenti che sono stati presentati.

Il Regolamento prevedeva e prevede che il Senato avrebbe dovuto consegnare, dopo 40 giorni complessivi, nella giornata di oggi - anzi il termine scadeva ieri sera - il complesso della manovra PRESIDENTE. Con l'accordo dei Capigruppo abbiamo stabilito la conclusione per questa sera, quindi nessuna obiezione. I tempi sono stati gestiti con una certa larghezza doverosa, visto che i lavori sono andati avanti molto ordinatamente. Ho l'obbligo di rispettare i tempi che abbiamo deciso assieme e, sia pure con quel minimo di elasticità che il senso di serietà consente,

cinque minuti per l'illustrazione dei subemendamenti e per il parere sulla proposta di stralcio avanzata dal senatore D'Onofrio. Darei i cinque minuti da ora, in modo che le motivazioni possano essere affrontate tutte quante. Fuori da questo, violeremmo il Regolamento, mettendoci in condizione di non poter adempiere ai nostri obblighi: prego i Gruppi di valutare con serietà questa mia riflessione.

una questione che nasce da una complicatissima vicenda della maggioranza. È questa, infatti, che tende a non rispettare il termine di oggi, per i suoi problemi interni: il relatore ieri ha presentato un emendamento; avevamo deciso di presentare subemendamenti (come abbiamo fatto); poi vi è stata una divergenza politica

Signor Presidente, vorrei cercare di parlare nei termini più sobri possibile: che lo dica un leghista forse è strano, ma comunque cercherò di farlo, perché la questione non mi pare banale.

Su questa base, abbiamo contingentato i tempi, stabilito la data del voto finale e lavorato esattamente con questa sintonia. Che cosa capita?

Presidente! Questo è inaccettabile. Se la maggioranza - e non l'opposizione - presenta un testo così rilevante dovrebbe essere lei a dire che, per la dignità del Senato, dobbiamo discutere e non votare come delle persone senza testa.

vi state accorgendo di cosa state votando? Avevo presentato con il mio Gruppo un emendamento che avrebbe posto fine allo scandalo per cui i boiardi (mi consenta questo termine, capisco capisco che è forte, ma ha una sua validità formale) del Ministero del tesoro si spartiscono gratifiche milionarie.

decine e decine di migliaia di euro, alla faccia dei lavoratori, di quelli che prendono 300 euro al mese di pensione minima. Dopo Dopo di che, nell'emendamento avete messo che i nani e le ballerine di Stato possono prendere anch'essi stipendi milionari. Il ministro Mastella è intervenuto: forse non lo sapete e quindi ve lo dico io, cari colleghi,

Delle due l'una: o pensiamo che facciamo un lavoro sbagliato e poco rilevante e quindi dobbiamo prendere meno dei dirigenti di Stato o, se il nostro lavoro, come io credo, nobile e molto importante, il nostro emolumento deve essere la misura cui commisurare tutti gli altri. Abbiamo presentato un emendamento che stabilisce questo principio perché vogliamo difendere il principio, assolutamente condivisibile, che deve esserci

alla sua capacità di mediazione - che ci troviamo di fronte, rispetto agli accordi della passata riunione dei Capigruppo, ad un'enorme novità con questo stravolgimento dell'articolo 91 "notturno". Soltanto adesso, avendo potuto approfondire di che cosa in realtà si tratta, abbiamo capito che stravolge in vari aspetti la nostra tradizione giuridica, andando incontro, da una parte, alle esigenze degli amici degli amici, come hanno detto i Capigruppo che mi hanno preceduto, dall'altra, mettendo sul fuoco per demagogia quello che la pubblica opinione pensa, gonfiata da ciò che alcuni fino ad oggi ed in questi giorni hanno scritto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni, in base alle quali è a mio avviso ineccepibile la decisione preannunciata dal Presidente del Senato. Si è parlato di enorme novità: questo testo è stato votato in Commissione bilancio, era noto da tempo, con il parere favorevole del Governo. Quanto tempo è passato, Presidente?

rientra nel tetto onnicomprensivo. Se l'insegnante del Conservatorio con l'incarico rimane sotto il livello del primo presidente della Corte di Cassazione, potrà svolgere tale ulteriore attività. Quindi, raccomando un'attenta lettura del testo.

questa sia una misura non solo di moralizzazione, ma dello Stato di diritto. Presidente Castelli, non c'è alcuna retroattività della norma. Lei ha segnalato dei casi che effettivamente colpiscono, compresi quelli dei magistrati che lavorano al Ministero della giustizia, che, a volte, guadagnano il doppio rispetto al primo presidente della Corte di Cassazione. Benissimo, ci aiuti: voti la norma che impedirà per il futuro il ripetersi di tali scandali. Questa norma consente anche di risolvere il problema dai voi sollevato dei funzionari del Tesoro che si spartiscono i proventi dell'evasione fiscale; il Gruppo della Lega voti tale proposta e ciò non accadrà più. *(Applausi dai Presidente, vorrei far rilevare all'Aula a questo punto della discussione che quest'anno, per la prima volta nella storia dell'attività parlamentare repubblicana, il relatore ed il Governo sia in Commissione sia in Aula non hanno presentato alcun emendamento nuovo e che i pochissimi emendamenti presentati sono consistiti nella riformulazione o nella correzione dei testi degli articoli approvati in Commissione. Quindi l'attività espletata è stata rispettosissima dei tempi e delle decisioni unilateralmente assunte dalla Commissione. Secondo punto. Ieri sera, all'esito della discussione che c'è stata, in particolare

conterrebbe innovazioni diffuse e radicali. Ho già detto in sintesi stamattina che così non è, perché la prima parte, il comma 2 di tale testo, non contiene alcuna modifica sostanziale, né rispetto al testo dell'emendamento di ieri, né rispetto al testo votato dalla Commissione. In particolare, si conferma il limite a regime per tutti i soggetti indicati nella norma della retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione, con alcune eccezioni che sono esattamente individuate in tutti e tre i testi (quello della Commissione, quello di ieri e quello di questa mattina), ovvero per le attività professionali ed i contratti d'opera per le società che hanno necessità di competere sul mercato in condizioni di efficienza, per le Autorità indipendenti e la Banca d'Italia, per le società quotate e per le 25 unità rimesse al Governo. Quindi, a regime,

ed una graduazione della decurtazione per gli altri contratti, quelli di diritto pubblico, per i quali si conferma questa decurtazione graduale, quadriennale, del 25 Questo è tutto, signor Presidente, onorevoli colleghi: io non capisco dove sia lo stravolgimento del testo e della norma. Approfitto, e concludo, per comunicare per comunicare all'Aula che ho presentato un subemendamento come relatore che contiene alcuni aggiustamenti di *drafting* irrilevanti (richiami di commi ed articoli) ed una rettifica resasi resasi necessaria in virtù di un errore materiale, nel senso che vi era una differenza tra il testo coordinato ed il testo dell'emendamento presentato. Nel testo dell'emendamento si faceva riferimento, a proposito del regime transitorio, ai rapporti in corso; nel testo coordinato dell'articolo si faceva riferimento invece ai contratti di diritto privato in corso. Si è provveduto ad adeguare il testo dell'emendamento rispetto al contenuto, che era quello voluto,

sui rimanenti articoli ed emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria. La seduta proseguirà ad oltranza, senza orario di chiusura prestabilito. La discussione riprenderà ora dall'articolo 92. L'articolo 91, nel nuovo testo proposto dal relatore, e i relativi subemendamenti saranno trattati per ultimi, dopo gli ulteriori articoli ed emendamenti precedentemente accantonati. Ai Gruppi di opposizione e al Gruppo Misto, che hanno esaurito i propri tempi, sono attribuiti ulteriori 30 minuti ciascuno per la discussione dei residui articoli ed emendamenti, escluse le dichiarazioni di voto finali. I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30 per le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge finanziaria. Dopo il voto con la presenza del numero legale, avranno luogo l'informativa del Governo sull'uccisione di Gabriele Sandri e i successivi incidenti e i relativi interventi dei Gruppi. Sempre nella giornata di domani, saranno votati la Nota di variazioni al bilancio, non appena presentata dal Governo, e il disegno di legge di bilancio nel suo complesso (anche quest'ultimo voto con la presenza del numero legale).

è la prima volta, in questa legislatura, che viene approvato un calendario a maggioranza. Ce ne dispiace. Prendiamo atto, signor Presidente, che ella non ha tenuto conto della proposta formulata in Conferenza dei Capigruppo da parte dell'intera opposizione, cioè quella di consentire all'Aula di esitare questo provvedimento entro la settimana. Abbiamo spiegato

In un anno e mezzo di percorso parlamentare, abbiamo riconosciuto in lei un grande mediatore,

Credo non sia mai successo nella storia del Senato che si presentassero così pochi emendamenti alla manovra finanziaria. Del resto, resto, ci eravamo dati delle regole perché volevamo un confronto a parità di condizioni, volevamo cioè discutere, proporre, emendare, votare. Ma questa parità di condizioni doveva essere rispettata dalla maggioranza e dal Governo, che invece, tutte le volte che si sono trovati in difficoltà, hanno deciso di buttare la palla al di là del campo, chiedendo accantonamenti e prendendo tempo.

le regole vanno rispettate da entrambe le parti, devono essere paritarie. Le modalità di comportamento devono obbedire a principi identici. Noi li abbiamo rispettati, la maggioranza e il Governo fino a ieri sera. Infatti, in presenza dell'intervento del Ministro della giustizia che poneva alla sua maggioranza e al Governo del quale fa parte

Allora ci si trova dinanzi a nuovi emendamenti, a richieste di possibilità di emendare entro un'ora testi complessi ed articolati,

Questo è lo scenario, signor Presidente, uno scenario che ho delineato in piena coscienza e consapevolezza. A me spiace che un Capogruppo della maggioranza si sia lasciato andare a dichiarazioni che - secondo me - non si attagliano al ruolo di Capigruppo che ricopriamo. Caro collega Russo Spena, io non prendo ordini da nessuno: prendo ordini dalla mia coscienza e nessuno mi ha ordinato di fare ammuina! Faccia ammenda delle sue espressioni,

a certe espressioni come altre che abbiamo ascoltato recentemente in Conferenza dei Capigruppo, dove un'altra Capogruppo dell'estrema sinistra si è permessa di offendere l'opposizione sostenendo che noi, chiedendo l'intervento del Governo e la possibilità

*FI)*. Signor Presidente, non ci stiamo - è la prima volta che succede - a questo andazzo. Non ci stiamo perché riteniamo che sia sacrosanto diritto dell'opposizione, di questa opposizione, della quale sono fiero di far parte assieme ai Capigruppo

perché la norma di questa mattina è un'intera legge, non è un articolo o un emendamento. Noi intendiamo intervenire sul tema del calmieramento dei costi dei *manager* pubblici. Non intendiamo sottrarci, ma intendiamo farlo con coscienza, con consapevolezza e con responsabilità. Nessuno sino ad oggi può arrogarsi il diritto di dire che questa opposizione in tale percorso non ha avuto responsabilità, consapevolezza e serietà. E proprio perché forti di questo nostro atteggiamento, forti di questa nostra consapevolezza, forti del fatto che il Paese guarda a noi, a quello che fa l'opposizione in Senato, forti di questa circostanza, io io contesto questo calendario e propongo personalmente quanto ho detto nella Conferenza dei Capigruppo: finire i lavori entro la giornata di venerdì per fare in modo che si discuta seriamente e serenamente su tutto il resto, perché ci sarà da discutere.

credo che questi fatti debbano obbligatoriamente farci riflettere su quanto politicamente si sta determinando in questa fase conclusiva della discussione della finanziaria e della legge di bilancio. Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale è rammaricata che non si sia giunti alla definizione di un calendario condiviso; e metodo, del resto, che da un anno e mezzo puntualmente si determina in tutte le Conferenze dei Capigruppo. Perché non si arriva a questo? Credo che il motivo fondamentale sia legato proprio al contrasto che c'è all'interno della maggioranza, perché quando un Presidente (e cioè lei, presidente Marini), che ha dimostrato ampiamente di essere capace di sintesi e di mediazioni alte, in una fase come questa di conclusione, come prima dicevo, a trovare una sintesi, significa che è fortemente condizionato dai contrasti che ci sono all'interno degli schieramenti di maggioranza. Questo è palese perché, come veniva prima detto nell'intervento del collega capogruppo di Forza Italia, senatore Schifani, noi non vogliamo assolutamente creare elementi tali da far saltare un impegno che questo ramo del Parlamento ha preso nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, cioè quello di licenziare il provvedimento entro il 16 di questo mese. Noi ci siamo attenuti scrupolosamente a questo percorso

l'introduzione di una nuova norma nella discussione della finanziaria, elementi tali da indurci ad approfondire e quindi a concorrere al lavoro, svolgendo appieno il nostro ruolo

nei confronti della sintesi, elementi tali da migliorare i provvedimenti. A fronte di ciò, noi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto di discutere di più, di più, di approfondire di più, di capire meglio che cosa è accaduto da ieri sera, perché non possiamo assolutamente sottovalutare la presa di posizione di un Ministro di questo Governo, del ministro Mastella, che dal banco del Governo - sottolineo: dal banco del Governo - è intervenuto in qualità, non solo di senatore, ma direi anche di segretario del suo partito, dicendo chiaramente: l'articolo 91 io non lo voto, l'articolo 91 non deve passare, l'articolo 91 rappresenta un *vulnus* nel percorso di questo provvedimento. Sembra che si voglia sottovalutare quanto è stato fatto e quanto è stato detto.

Se ci sono problemi nella maggioranza, che ancora una volta sono stati dimostrati e ampiamente conclamati, lei, signor Presidente, deve dare la possibilità a chi vuole lavorare,

l'opposizione ha mostrato, proprio in questo momento, in queste giornate, in queste settimane di sessione di bilancio, il massimo della responsabilità.

in Aula, quando i nostri emendamenti sono stati ridotti a qualche centinaio e, nel corso dei lavori, molti sono stati anche ritirati, a documentazione della trasparenza del nostro messaggio politico e, quindi, della nostra volontà politica. Non comprendiamo, signor Presidente, la reazione da parte della maggioranza maggioranza e i motivi per i quali si vuole strozzare un dibattito così importante ed impegnativo anche sull'emendamento (che emendamento non è, ma è ben altro) che il relatore ha presentato ieri sera e riformulato questa mattina. Nella lettura dei due emendamenti, il primo e il secondo, si dimostra ampiamente che si

non per arrivare a risultati politici, ma ad una mediazione che è stata solo e soltanto una trattativa per poter riequilibrare una frattura. E la trattativa non è stata su argomenti che possono rappresentare luci all'interno dell'Aula ma è stata una trattativa clientelare, solo e soltanto tale, per fare in modo che si rimettessero insieme

come mi sembra si voglia fare, attesa la soluzione emersa dalla Conferenza dei Capigruppo, credo che daremmo uno spettacolo negativo, ancor più in queste ultime ore di dibattito sulla finanziaria.

Sono convinto che verrà illuminato nel corso dei lavori perché, conoscendola, anche per quanto ha dimostrato e dimostra continuamente, lei non condivide questa scelta, non può condividerla. Ci auguriamo, Presidente, che si possa effettivamente, serenamente riunirsi, definire i tempi, far sì che si abbia la possibilità di stare anche una giornata in più nel discutere e dibattere di questi argomenti e arrivare serenamente ad un voto che l'opposizione ha voluto; un voto libero e non condizionato

Basta ditelo a voi stessi, perché chi dice «basta» significa che non ha né idee da proporre né capacità per capirle ed ascoltarle

dell'emendamento presentato questa mattina dal relatore dopo la sospensione di ieri sera, di avere più tempo di riflessione e anche di discussione in Aula. Questa è stata la ragione per cui, assegnando un tempo ulteriore ai Gruppi che l'avevano esaurito, ho proposto di spostare la conclusione dei nostri lavori, che dieci-quindici giorni fa i Capigruppo, assieme con me, avevano fissato per la giornata di mercoledì, a domani, dando un tempo di approfondimento, riflessione e intervento anche su quel punto. Oltre questa possibilità non possiamo andare, perché diventa un fatto politico per il Senato spostare, non di quel congruo tempo che la complessità dei nostri dibattiti comporta ma sensibilmente, i termini della conclusione dei nostri lavori. Questa è la mia preoccupazione, legata solo

Noi siamo il Senato che aveva deciso parecchi giorni fa di concludere le votazioni sulla finanziaria entro oggi. Perché stiamo discutendo dell'eventualità di andare oltre questo termine, di andare oltre un tempo congruo,

di ottenere un risultato che è del tutto compatibile con l'approvazione della finanziaria in tempo utile, ragionevolmente entro Natale, da parte delle due Camere. Non stiamo chiedendo di non la finanziaria e di andare all'esercizio provvisorio; se avessimo posto tale questione avrei capito se da parte della maggioranza si fosse detto: «No, non possiamo accettarlo». Noi stiamo chiedendo una una revisione, come avvenuto con la proposta del nuovo calendario da parte del Presidente del Senato, che preveda una prosecuzione dei lavori la cui conclusione era stabilita per oggi. Per quale ragione? Per un capriccio dell'opposizione? Perché vogliamo perdere tempo? Perché non sappiamo cosa fare domani? Perché qualche giornale dice che alcuni colleghi senatori domani potrebbero non esserci? Nessuna di queste ragioni, perché i senatori che potevano non esserci hanno opportunamente dichiarato che ci saranno anche domani e penso dopodomani. Se non ci sono fatti strumentali, c'è un fatto assolutamente ragionevole.

riflettesse un attimo in più. È stato detto dal collega presidente Salvi e da altri della maggioranza che il famoso articolo 91 della finanziaria, quello che modifica radicalmente il sistema di diritto di diritto privato e di diritto pubblico relativo a tutti gli incarichi nella pubblica amministrazione (si tratta cioè di una rivoluzione totale), è fondamentale per la finanziaria. Il ministro Mastella ieri ha detto che non lo avrebbe votato. Ora, delle due l'una: o ha parlato come Ministro della giustizia, preoccupato di problemi di ordine giurisdizionale,

o il ministro Mastella era contrario all'ispirazione di fondo della finanziaria, che trovava in questo articolo un punto determinante della propria manovra, e allora era fuori della maggioranza politica. Ecco perché ho chiesto al relatore a nome di chi il senatore Mastella aveva parlato. Di questo problema politico volevamo discutere con adeguatezza, per capire se il nuovo testo che il relatore ci ha presentato stamattina ha risolto i problemi di tipo giurisdizionale, soprattutto quelli relativi alla tutela dei dritti dei cittadini, in quanto il ministro Mastella aveva parlato come Ministro della giustizia, oppure se ha risolto i problemi politici in quanto quell'articolo, non essendo neanche lontanamente provvisto di copertura, non era decisivo per la finanziaria. Per queste ragioni ho presentato, come Capogruppo dell'UDC, la proposta di stralcio, perché lo stralcio presuppone che nel merito l'argomento debba essere trattato ma che probabilmente può non essere decisivo per la finanziaria. Se il ministro Mastella ieri ha parlato da Ministro della giustizia,

Ho pensato che, evidentemente, il ministro Mastella avesse parlato in dissenso radicale nei confronti del provvedimento, e questo poneva un problema di maggioranza politica e di contenuto, da cui lo stralcio. Non mi si può dire che c'è l'intenzione di giocare sugli argomenti. Ancora adesso non abbiamo capito quali sono le ragioni di ordine giuridico per le quali il ministro Mastella ha parlato contro il testo del relatore di ieri e quali sono le novità del testo di oggi. Abbiamo diritto di discutere per 24 ore di queste cose e quindi di votare la finanziaria venerdì e non domani, o chiediamo cose impossibili? Votare la finanziaria venerdì significa rendere impossibile la finanziaria entro l'anno? No,

Se si fosse deciso che si sarebbe votato alla Camera venerdì mattina avrei capito che la nostra proposta era contraddittoria con il sistema bicamerale, ma così non è. La ragione di fondo per la quale il collega Schifani prima ha rilevato una circostanza della quale mi permetto di

che il Senato è chiamato a discutere di un calendario approvato non all'unanimità. Ci si rende conto che nel Senato della Repubblica non sarebbe possibile, non dico fare molte cose, ma proprio nulla se non vi fosse un minimo di consenso almeno sul calendario? Ci si rende conto che il dissenso sul calendario concorre a rendere impossibile il funzionamento procedurale del Senato della Repubblica? Allora perché il Presidente del Senato è indotto

può approvare il calendario anche contro l'opposizione (non è una novità), ma lo fa soltanto in una logica di guerra guerreggiata. Se la maggioranza vuole la guerra guerreggiata nei confronti dell'opposizione non può lamentarsi che guerra guerreggiata ci sia. È il Presidente del Senato che viene in discussione come Presidente di un'Assemblea nella quale si svolge una guerra politica tra due componenti e dove non esiste più l'organo superiore che dovrebbe essere il Presidente del Senato. Ecco perché la nostra richiesta di andare entro questa settimana, è compatibile con la votazione della finanziaria da parte di entrambe le Camere nei tempi utili, ed è del tutto compatibile con i tempi che la Camera ha stabilito per votarla, nonché con i problemi che sono stati posti non da noi ma ieri nel corso che poteva essere valutato politicamente, e lo faremo a parte, tra il ministro Mastella e il relatore. Non abbiamo capito se lo scontro ineriva alla tutela dei diritti, perché il nuovo testo non dà garanzie - ma, ripeto, ne parleremo nel merito - o invece era un'opposizione al principio di avere questa questa novità all'interno della finanziaria; da qui la proposta di stralcio. Ancora un'ultima preghiera, signor Presidente. Nell'interesse dell'istituzione che ella presiede, non dia vita per la prima volta alla presa d'atto che c'è una guerra civile in quest'Aula, dove c'è soltanto la volontà di lavorare nell'interesse del Paese

e, almeno per quanto riguarda me, conosco le difficoltà legate all'approvazione del calendario in Aula. Ma per un anno e mezzo questo lavoro è stato svolto con grande determinazione

dai colleghi che mi hanno preceduto, e cioè di arrivare a venerdì, se ciò risultasse necessario. Ma vorrei articolare le motivazioni per cui mi sento di sostenere tale proposta. Devo darle atto, Presidente, che lei in questo anno e mezzo ha vigilato con grandissima attenzione sul fatto che il dibattito non dovesse essere in nessun modo conculcato. Su questo non c'è il minimo dubbio, tanto è vero -

Mi richiamo proprio a questa sua capacità di cercare sempre di comprendere le questioni da un punto di vista oggettivo, mai ricordandosi da quale parte politica proviene, per formulare questa mia proposta. Lei dice che è un impegno politico

Abbiamo discusso sempre e comunque nel merito della legge, non abbiamo mai fatto ostruzionismo e ci siamo autolimitati ulteriormente con gli emendamenti. Senatore Boccia, lei non può dirci lei non può dirci che abbiamo disatteso gli accordi perché avevamo promesso di tagliare un certo numero di emendamenti e poi ne abbiamo tagliato qualcuno in meno. Di fatto, l'autolimitazione è del tutto evidente.

perché ci si propone di arrivare al voto domani e noi proponiamo di arrivarci dopodomani, possibilmente in mattinata. La differenza è ormai molto piccola; è piccola dal punto di vista cronologico ma non lo è dal punto di vista sostanziale. Per quale motivo? Colleghi, non vorrei diventare retorico e dire cose esagerate, però non c'è il minimo dubbio che questa disgraziata seconda Repubblica ha avuto un comune denominatore, cioè la debolezza della politica. Noi siamo deboli, ma siamo stati tutti succubi della magistratura, siamo succubi dell'alta burocrazia dello Stato, che fa ciò che vuole. Chi è stato al Governo sa che non c'è verso in alcun modo di prendere giuste decisioni contro l'alta burocrazia, perché si coalizzano, perché poi arriva la telefonatina dal Quirinale che ti minaccia - più o meno velatamente - che non ti sarà firmata la legge se inserirai quella norma, e allora devi toglierla. Bene, siamo arrivati a un punto in cui forse la politica sta rialzando la testa, ciascuno dal proprio punto di vista. Non vorrei affermare qualcosa di straordinario, ma se se riusciremo a recuperare il ruolo della politica, forse passeremo dalla seconda, magari se non alla terza, alla seconda Repubblica e mezzo. Questo è uno snodo cruciale della nostra vita politica e parlamentare. Possiamo avere il tempo di discuterne oppure no? O dobbiamo essere banalmente legati ai trenta minuti perché in finanziaria si presenta l'emendamento per il finanziamento della chiesa di Roccacannuccia? Non stiamo discutendo di quello. Ripeto, siamo arrivati a uno snodo fondamentale della nostra vita istituzionale

Vogliamo ritornare al primato della politica sì o no? Con questi emendamenti ciascuno per la propria parte sta tentando di compiere questo percorso.

e vi chiedo se vi sembra il caso - solo per poter dire: abbiamo votato domani sera, anziché venerdì mattina. Pongo semplicemente tale problema, soprattutto a coloro i quali hanno anche scritto libri su tali questioni, sui costi della politica, sul ruolo dei parlamentari rispetto alla burocrazia, sugli sprechi del Paese. Vogliamo essere conseguenti anche in quest'Aula oppure deve sempre prevalere una strana ragion di Stato?

non so se ci sono dei precedenti: sicuramente non ve ne sono nella scorsa legislatura. Vorrei ricordare che lei ha concesso 30 minuti a ciascun Gruppo dell'opposizione,

ieri, alle 14, i tempi erano esauriti. Quindi i tempi di ieri pomeriggio e di questa mattina sono già aggiuntivi.

Regolamento. Noi ci associamo a questa richiesta e ci auguriamo di poter continuare i nostri lavori, in maniera che, nel rispetto del Regolamento, si possano sviluppare le azioni dell'opposizione

Nella proposta fatta dal Presidente c'è la continuazione dei lavori fino all'esaurimento della discussione degli articoli e degli emendamenti.

intervenire per poter spiegare esaustivamente le motivazioni che lo portano a chiedere una modifica del calendario, e non credo che questa esigenza possa essere soddisfatta in due minuti. Presidente Schifani, l'armonizzazione è un dovere del Presidente, quando ci sono obiettivi che sono presenti all'Assemblea. Io rispetto la libertà del parlamentare

per spiegare le ragioni della difformità del nostro parere in relazione all'andamento dei lavori in quest'Aula e soprattutto alla fissazione del calendario, che poi inevitabilmente sarà messo ai voti dell'Aula, in quanto per la prima volta in Conferenza dei Capigruppo non ci siamo trovati d'accordo su una medesima scadenza. Midispiace che il collega Boccia abbia detto le cose che ha detto, ma le comprendo, nel senso che fa il suo dovere come portavoce della maggioranza quando si tratta di difendere i lavori d'Aula, pure quando questi però, collega Boccia, hanno avuto le forzature che hanno avuto. Già questa mattina sono intervenuto asserendo che è vero che il comportamento della Presidente del Senato, come sempre, è stato correttissimo, nel quadro dell'accordo che avevamo raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo. È la maggioranza, con le sue divisioni, che ha cambiato quell'accordo e l'andamento dei tempi nell'Aula: abbiamo dovuto interrompere più volte, anche per errori materiali del Governo in relazione alle coperture della finanziaria,

quindi siamo nella nostra capacità e possibilità politica di argomentare. Con la novità dell'articolo 91, stravolto, come ho dimostrato in Conferenza dei Capigruppo a qualcuno più incredulo, perlomeno per il 50 per cento della sua prima stesura, è di tutta evidenza che non ci troviamo più di fronte ad un articolo, ma ad una vera e propria legge nuova,

sui 25 è uno degli elementi più evidenti di partigianeria o di preparazione di qualche cosa che ancora non abbiamo compreso nel suo peso politico ed amministrativo e vorremmo avere il tempo di poterlo approfondire.

contenuta nell'articolo 91, per cui ci piacerebbe portarle avanti insieme. Vorremmo incardinare anche quel provvedimento all'interno del calendario da noi previsto fino alle ore 21 di venerdì.

nei cinque anni della scorsa legislatura, quando noi eravamo opposizione, cercando di contemperare le esigenze legittime dell'attuale opposizione con le esigenze di governare i processi, i procedimenti, le votazioni che in quest'Aula si svolgono. Signor Presidente,

tutte aventi una priorità particolare. No, noi parliamo di una Conferenza dei Capigruppo che aveva un unico oggetto, un unico disegno di legge e, rispetto a questo disegno di legge finanziaria, i limiti di discussione. proprio perché a monte l'oggetto della discussione era limitato, si comprende benissimo che anche a valle dovrà essere per forza limitato.

oggi potrebbe far comodo a voi, domani a noi. Noi invece abbiamo a cuore il rispetto di quelle regole, anche non scritte, che devono certificare l'agibilità democratica delle istituzioni. Oltre quel limite, colleghi, nessuno di noi può assolutamente andare. Ecco perché, Presidente, visto che lei ha già consentito ai Capigruppo di illustrare complessivamente le proposte - e quasi tutti i Gruppi lo hanno fatto - e che i limiti della discussione sono modesti, quando termina la discussione, oggi, venerdì o in qualche altro giorno, pure l'armonizzazione dovrà tener conto di questa limitazione obiettiva. Altrimenti entreremmo in un arbitrio che testimonierebbe una volontà che non esiste, cioè quella di un atteggiamento ostruzionistico defatigatorio, che fin qui onestamente non c'è stato, se è vero, come è vero, che in Commissione avete consentito che si andasse avanti nei lavori e che ordinatamente siamo arrivati fino alla fine del provvedimento. Però è chiaro che le singole situazioni vanno verificate e i limiti oggettivi delle valutazioni che oggi il Regolamento affida alla Presidenza sono, secondo me, abbastanza precisi. In questa logica,

si sono contrapposte due proposte, il Regolamento non prevede che si possa ridiscutere di tutti i possibili calendari che si che si possono proporre, ma solo che si pongano in ballottaggio la proposta prevalente e quella soccombente. Questo non è scritto da nessuna parte, parte, perché il nostro Regolamento ha una forza compulsiva sull'Assemblea nel momento in cui l'unanimità della Conferenza dei Capigruppo stabilisce l'accordo e impedisce a ogni senatore financo di formulare proposte: ossia, se il mio presidente di Gruppo ha negoziato un accordo in sede di Conferenza dei Capigruppo io non posso

e nel momento in cui la parola passa all'Assemblea la facoltà di proposta, secondo il Regolamento, non è più in capo ai Gruppi, ma ai singoli parlamentari,

per avere acquisito agli atti l'emendamento che era stato presentato con lieve ritardo rispetto alla scadenza. Per quanto riguarda il calendario, signor Presidente, lei ha detto che il calendario vigente è quello che prevedeva la chiusura dei lavori questa sera e vi è il problema di aggiustare i tempi.

Siamo di fronte a questo testo che ci è pervenuto stamattina, con una guerra civile interna alla maggioranza...

Presidente, spero di poter parlare al Presidente e non ad una fotocopia. Francamente, se lei avesse cercato la mediazione nella Conferenza dei Capigruppo non ci sarebbe stata questa serie di interventi, i fatti si producono con gli atteggiamenti. Vorrei, possibilmente con i tempi che lei ha concesso al senatore Manzione, riportare il discorso, proprio usando i suoi temi, su una proposta che riguarda esattamente il calendario che lei ci ha letto. Vede, Presidente, non voglio utilizzare questo tempo per replicare ad altri colleghi. Semplicemente mi è dispiaciuto quello che ci ha detto il collega Antonio Boccia. Ha trovato un'opposizione disponibilissima durante questa finanziaria e ci viene a dire che ci fanno la carità di qualche minuto in più. Il collega Boccia riservi la carità a quelli per i quali stanno preparando gli emendamenti di notte e di giorno. Ma voglio andare alla proposta, perché il Presidente ci ha chiesto di attenerci al tema. Voglio che l'Aula valuti la possibilità di andare oltre il termine proposto di venerdì, Presidente (esattamente come ci dice il senatore Manzione, nei limiti della proposta emersa nella Conferenza dei Capigruppo), ha il dovere di farci discutere di tre questioni che riguardano esattamente quanto è previsto nel calendario dei lavori. La prima questione è evidente: è la legge finanziaria. Credo, Presidente, che sia molto parsimonioso il suo atteggiamento nel concedere 30 minuti a ciascuno dei Gruppi che intende intervenire, quando allo stato 40 subemendamenti e ce ne saranno altri del relatore sugli emendamenti accantonati. Avremo il diritto e la possibilità di presentare altri subemendamenti. Mi dica lei se questo è un percorso che può essere accettato. La seconda questione, Presidente, è collegata alla legge finanziaria. Ieri sera l'opposizione...

La seconda questione riguarda l'intervento del ministro Mastella di ieri. Non abbiamo chiesto un dibattito su quello che è un fatto nuovo, rappresentato dalle dalle comunicazioni del ministro Mastella. Non ho dimenticato - e il Resoconto stenografico è qui a raccontarcelo - che il senatore Salvi ha chiesto al ministro Mastella a che titolo parlasse.

Abbiamo il diritto di sapere se il ministro Mastella ha posto questioni vere e serie sull'emendamento originario e quali sono, perché si è trovato l'accordo e su che cosa. Credo sia una questione importante. La terza questione, Presidente, è in certo senso più delicata.

La terza questione riguarda l'argomento portato qui in Aula, ossia l'informativa del Ministro dell'interno sulle questioni riguardanti i drammatici fatti in cui ha perso la vita un giovane tifoso. Presidente, possiamo chiedere, ai fini del calendario dell'Aula, che quel dibattito non si limiti ad un'informativa, ma che ci sia la possibilità di presentare proposte di risoluzione e di avviare una discussione su quello che è successo? È possibile inserire

di poter lavorare anche sabato se occorre, non obbligatoriamente, per avere la possibilità di discutere seriamente anche sulla informativa del ministro Amato con il voto dell'Aula.

Ha una sua logica in presenza di una scadenza di decreti‑legge, di norme che vanno approvate inderogabilmente entro una certa data, pena la loro decadenza. Ha una logica in presenza di un calendario complessivo dei lavori d'Aula che vedrebbe l'Aula impegnata per altri temi, per decreti-legge in arrivo, quindi in relazione ad effettive, articolate ed obiettive motivazioni che impongono alla Presidenza di disciplinare i lavori in quanto i lavori di Aula sono obiettivamente compressi da una molteplicità di temi.

addirittura la possibilità di lasciare libera l'Aula la prossima settimana perché mancano dei provvedimenti che hanno una concreta urgenza di esame.

Questo è il ragionamento che faccio, perché ha detto bene il collega Manzione quando ha richiamato la norma da lei citata sull'esigenza di armonizzazione dei tempi tempi e applicata molto opportunamente dal presidente Pera nella precedente legislatura. Però, signor Presidente, mi consenta di dire che nella precedente legislatura c'era un Governo che legiferava, che faceva arrivare i provvedimenti in Parlamento, che decretava

l'eventuale utilizzazione di questa norma regolamentare. Non vorrei, infatti, che le si possa muovere la contestazione di essersi avvalso di questa norma in assenza dei presupposti che postulavano

Schifani, il suo richiamo l'ho ben presente. Il Regolamento stabilisce i tempi nei quali dobbiamo trasmettere all'altra Camera il testo e a ragione di un lavoro che non si esaurisce nell'Aula, ma nelle Commissioni.

una proposta diversa. D'ALI' *(FI)*. Signor Presidente, con buona pace di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, penso di essere uno tra coloro che hanno la maggiore consuetudine con quest'Aula (non con l'attività parlamentare) in ragione della mia permanenza in Senato. Nella mia memoria vi è sempre un

e di poterlo fare anche con riferimento ad alcuni emendamenti che sono stati accantonati - penso a quello, importantissimo, sui talassemici - e che, non ancora risolti perché il Governo non ci ha dato le indicazioni necessarie

Abbiamo, tra l'altro, oltre ai vari accantonamenti, l'articolo 91. Nato dal Governo, con una norma di una colonna del testo stampato, in Commissione è diventato un testo di sei colonne;

norma non dovesse avere effetto retroattivo in realtà è disattesa, perché la norma ha effetto retroattivo. Vogliamo avere il tempo e il modo di spiegarla, di approfondita e di capire dove vuole arrivare

per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute». Presentato lo scorso gennaio, dopo un approfondito dibattimento in Commissione, il provvedimento è in attesa della sua calendarizzazione in Assemblea. La mia volontà di intervenire in Aula oggi discende dalla consapevolezza mia e di tutti i miei colleghi dell'importanza del provvedimento suddetto e, soprattutto, dell'importanza di una sua calendarizzazione immediata in Aula al fine di aprire un dibattito serio e costruttivo su un tema complesso come quello della semplificazione amministrativa in materia di salute, che ricomprende le misure volte a garantire l'efficienza del Servizio sanitario nazionale,

la proposta avanzata dall'opposizione di avere più tempo a disposizione. Non si può affrontare un argomento così delicato come quello previsto dall'articolo 91 della legge finanziaria con mezz'ora di tempo, quando si va toccare tutto l'apparato dello Stato. Noi vogliamo sapere come si è arrivati a questo numero di 25 persone, i super-*top*. Vogliamo sapere come mai il ministro Mastella ha cambiato opinione rispetto alla posizione espressa ieri sera, allorquando ha determinato una rottura nella maggioranza con le modifiche che riguardavano il problema dei compensi e delle prestazioni professionali della RAI, compreso quello dell'amico Santoro, che viene salvaguardato da questa norma. la mia proposta è molto semplice. Le chiedo, per rispettare i termini della sessione di bilancio, che si vada ad oltranza, anche con seduta notturna,

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, queste nostre eccezioni non sono sicuramente strumentali: le sta rendendo tali lei per opporsi a

Lei, Presidente, non ha fatto una proposta di armonizzazione, che comunque avrebbe dovuto essere votata dall'Aula e non essere da lei imposta. Lei sta proponendo una normalizzazione, probabilmente suggerita da qualche rivoluzionario di ottobre della sua parte politica a sinistra. a sinistra. Noi abbiamo di fronte l'articolo 91 della finanziaria che cambia alla radice l'ordinamento, perché modifica i contratti nazionali di lavoro dei dirigenti, dei dirigenti, i rapporti sindacali all'interno della pubblica amministrazione e fa cadere il libero gioco della domanda e dell'offerta, quindi della concorrenza

La seduta è ripresa. Comunico all'Assemblea l'organizzazione dei nostri lavori come stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo con decisione unanime. Questa sera riprendiamo subito i lavori e la durata della seduta sarà fino alle ore 21. Domani, giovedì, sono previste due sedute:

al Gruppo Misto, escluse le dichiarazioni di voto finali.

Presidente, dall'inizio della seduta, ho tentato disperatamente, come possono confermare gli Uffici, di prendere la parola. In questa parola. In questa legislatura, anche i Presidenti di Commissione stanno attuando una specie di eversione regolamentare

presentato dal senatore Villone in Commissione bilancio, con il quale si prevedeva il taglio della dotazione degli organi costituzionali. L'inammissibilità di questo emendamento traeva origine da una normativa che vieta l'invasione delle prerogative degli organi costituzionali.

Fu obiettato dal sapiente Presidente della Commissione bilancio che questo emendamento doveva essere ammesso quindi contraddicendo gli Uffici - secondo parametri di natura politica. Questa gravissima affermazione

sapere se gli interventi di qualsiasi genere sono ricompresi nel tempo messo a disposizione e se, una volta esauriti i tempi, sono previste o meno proroghe.

proposta al Governo e naturalmente anche alle concezioni economiche e politiche della destra. Credevo e credo che, dopo l'iniqua manovra dello scorso anno, fosse necessario intervenire contro i privilegi fiscali permanenti alle imprese e ridurre fortemente le spese militari per risarcire i lavoratori e le classi più deboli. Non è stato così. Non è così, anzi. Prendo atto che questo mio tentativo non ha avuto successo che i miei emendamenti fondamentali sono stati respinti dalla maggioranza a rigetto di una vera stabilizzazione del lavoro precario (che avrà un colpo mortale con il Protocollo sul *welfare*), a rigetto del recupero del *fiscal drag* della tassazione delle rendite; per non dire del finanziamento dei CPT, del Vertice del G8 in Sardegna e persino del mantenimento dei privilegi fiscali alla Chiesa, dando un ulteriore grave colpo alla laicità dello Stato. La mia posizione politica, quindi, è molto netta. Sono all'opposizione da sinistra a questo Governo e a questa maggioranza. Naturalmente sono più che mai distante dall'opposizione di destra.

considero esaurita la mia battaglia su questa finanziaria e abbandono il prosieguo dei lavori dell'Aula e dei voti naturalmente sulla finanziaria stessa. È compito di chi condivide questa politica garantire questa maggioranza. Non è il mio caso.

che vorrei permettermi di segnalare alla sua attenzione - è giusto il richiamo del senatore Boccia - è considerare quei 30 minuti nella quota dell'opposizione, perché altrimenti rischio di non avere possibilità di parlare.

o li sottopone a dei vincoli molto rigorosi per quanto riguarda, in particolare, un settore strategico quale quello dell'università e della ricerca. Credo sia questo un errore molto grave che rischia di costare caro al sistema universitario italiano, va in controtendenza rispetto

l'impiego privato. Con questo emendamento voglio avanzare una richiesta alle componenti veltroniane della maggioranza che, nelle scorse settimane, si sono dichiarate per un mercato del lavoro flessibile e per una pubblica amministrazione moderna. Credo che sia questo un banco di prova. Voi sapete che tutti i rettori delle università italiane si sono schierati pesantemente contro questo articolo della finanziaria, chiedendo che venisse quanto meno eliminato per il settore delle università.

che vuole un ritorno al passato su un tema così delicato. Voglio fare solo un cenno molto puntuale: la carriera d'ingresso dei

credo sia un vincolo molto stringente il non poter essere sostituiti da personale a tempo determinato, soprattutto di fronte a certe urgenze e necessità, che possono peraltro prolungarsi oltre ai famosi tre mesi. Quindi, chiedo la votazione elettronica e l'approvazione di questo emendamento. FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, la velocità con cui stiamo approcciando i lavori è probabilmente figlia

L'articolo 92, che si trova in mezzo tra il 91 e il 93 nella ferrea logica dei numeri, sembra di una importanza di secondo piano

sino al giorno 19. Allora, prendiamoci questo momento per ragionare sul comma 1 dell'articolo 92. Vede, Presidente: il comma 1 dell'articolo 92, facendo riferimento alla legge n. 165 del 2001, fa decidere all'Assemblea una disposizione per cui, se un giorno il ministro D'Alema volesse dismettere i panni del politico e dare un suo sì alla possibilità di essere chiamato alla consulenza di un'amministrazione particolare - non me ne voglia il ministro D'Alema, ma lo faccio per significare il ragionamento - non potrebbe farlo

il lavoro di consulente ad alcuno e ad alcunché, Presidente. Ma questa è, nell'organizzazione complessiva della finanziaria, un'altra prova specifica di come l'atteggiamento sia sia statalista, esclusivista, foriero di un complesso di disposizioni, ed evidentemente i colleghi non vogliono fare tesoro dei ragionamenti fatti da parecchi giorni in Aula.

che sta alla base degli emendamenti che presentiamo. Mi fa specie che su questa tipologia di emendamenti nessuno della maggioranza voglia intervenire: sono tutti laureati? Vogliono tutti continuare a fare i parlamentari? Nessuno vorrà fare da consulente ad alcuno e ad alcunché? Com'è possibile portare in secondo piano la discussione su una tipologia di disposizioni così gravi? È possibile che ad un dato momento si proponga tutto e il contrario di tutto a questa Aula e che comunque si sia perso il senso della ragione? Questa è una cosa cui non mi posso attenere, e non me ne voglia, Presidente, probabilmente perché, assieme ad altri colleghi, ho studiato così tanto la materia e non vorremmo che questa Aula proseguisse nei lavori commettendo errori su errori e approvando disposizioni che hanno un carattere assolutamente di diniego di quella che non è la buona sostanza ma il buono e giusto interesse dello Stato.

Presidente, la ringrazio di avermi richiamato alla calma, ma dall'altra parte dell'emiciclo si era sentito un coro di dissenso. Il coro di dissenso, se permette, lo richiamo anche perché è il motivo

quindi a questo punto ritengo che il Governo abbia la sicurezza di continuare a sopravvivere e che nessuno di loro vorrà fare il consulente ad alcuno e ad alcunché. Ma a questo punto ci sono gli emendamenti del relatore, per cui invece di

e il relatore propone la necessità di votare un emendamento che sostituisce la parola "e" con la parola "o", invece di voler rispondere a quelle che secondo me erano delle eccezioni che facevo al complesso della disposizione, che avevano tutta la loro valenza. Cioè, perdiamo tempo ad approvare un emendamento che sostituisce "o" con "e" e rivede "e" con "o", invece di dare una risposta a questa Aula. Questo il motivo per cui abbiamo chiesto di parlare, perché perlomeno quello che diciamo lo sente il Paese, visto che questa maggioranza e questo Governo sono sordi a tutte le buone ragioni.

Se non ho mal compreso, la Presidenza ha assegnato ai Gruppi di opposizione un ulteriore tempo di un'ora non con riferimento all'articolo 91, ma con riferimento all'intera finanziaria. È corretto? PRESIDENTE.

di rivedere il proprio parere negativo sull'emendamento che io propongo per queste ragioni: i commi 5 e 6 dell'articolo 92 prevedono, proprio per abbattere i costi e per contenere le spese, leggo testualmente: «l'attuazione di tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza». Il comma sesto prevede l'abbattimento del 10 per cento del tetto degli straordinari per l'intera pubblica amministrazione. L'emendamento riguarda il comma 8 perché, a differenza di ciò che è stato fatto altre volte in passato, le disposizioni dei commi 5 e 6 non sono escluse quanto ad applicazione per le Forze di polizia, per le Forze armate e per i Vigili del fuoco. Allora ho chiesto l'attenzione del Governo e del relatore perché vorrei sapere da loro come si esercita il lavoro a distanza per i Vigili del fuoco, cioè vorrei sapere, se tra le forme di lavoro a distanza c'è per esempio il telelavoro, come viene concretamente esercitato in funzione di ordine pubblico da parte delle Forze di polizia, o in esercitazioni da parte delle Forze armate. È evidente che questi due commi devono essere esclusi in quanto ad applicazione per queste categorie di lavoratori particolari, così come deve essere escluso il taglio degli straordinari del 10 per cento perché già oggi, come sanno tanti colleghi, qualunque sia il loro Gruppo di appartenenza e il loro schieramento politico, le le Forze di polizia arrivano a metà del mese e hanno esaurito il monte ore di straordinario per cui lo straordinario che si fa dopo si fa egualmente ma non viene pagato e quindi si lavora *gratis*, perché non c'è nessun operatore di polizia che mentre sta svolgendo un'attività di contrasto al terrorismo, ascoltando delle intercettazioni telefoniche di gruppi terroristici, o mentre sta inseguendo i partecipanti di una estorsione, si blocca perché è cessato il monte ore di straordinario. Ieri si è parlato, il Senato si è fermato per quasi 24 ore, di persone che in modo assolutamente legittimo raggiungono e superano tetti di reddito annuale di 300.000 euro. Qui stiamo parlando di persone che rischiano la vita per 1300 euro al mese. È indegno non votare un emendamento che moduli il taglio degli straordinari alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco e alle Forze armate.

sottolineando come l'articolo 92, che va letto in combinazione con l'articolo 93, contiene norme che apparentemente possono essere condivise, ma che poi estremizzano certe posizioni fino ad arrivare a conseguenze quali quelle che il collega Mantovano ha espresso in maniera molto chiara e che si cerca di evitare con l'approvazione di questo emendamento. Questo è un modo di operare tipico della maggioranza che ha usato in questi testi la clava, invece di usare il bisturi, e approvando queste norme senza questi emendamenti si rischia di causare un danno maggiore del beneficio che si vuole apportare alla pubblica amministrazione.

In questo modo prima abbiamo commesso un errore, ma capisco che non tutti gli emendamenti vengono letti. Adesso parliamo di un'altra questione. Si tratta dell'applicazione di quanto deciso già con la finanziaria dell'anno scorso e quindi della possibilità di realizzarlo. Spero che i colleghi abbiano letto l'emendamento che tenta di affrontare il problema dei lavoratori precari per gli enti locali

che noi dell'UDC abbiamo fatto della sicurezza una delle questioni strategiche, per un diverso profilo della finanziaria che abbiamo proposto sia come partito che come coalizione del centro‑destra.

sua preoccupazione, la paura che i cittadini di Roma e di tutta Italia stanno vivendo in questo momento e quindi le difficoltà che tutta

i numeri tragici di questa emergenza nel soccorso, nel presidio del territorio da parte della Polizia.

Soprattutto, come ricordava nell'emendamento precedente il collega Mantovano, sono bloccati gli straordinari. La Polizia che fa straordinari e festivi molte volte si trova a lavorare a credito o gratis verso lo Stato, proprio per il senso del dovere che ha. Ci troviamo di fronte - lo ha denunciato il ministro Amato - a una serie di procedure di sfratto delle caserme

Mi auguro che l'emendamento 95.3 venga finanziato proprio perché tutti insieme dobbiamo fronteggiare questa emergenza. Abbiamo anche presentato un altro emendamento, il 93.5, perché ci siamo fatti carico anche della carenza di personale di personale L'emendamento propone l'assunzione di 4.500 agenti, equamente distribuiti tra Guardia di finanza, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria e Polizia di Stato perché di fronte ai 10.000 pensionamenti che si registreranno nel triennio lo Stato propone che ne vengano riassunti soltanto 3.500. I responsabili dell'Interforze, che hanno tenuto una conferenza stampa due settimane fa, alla quale ha partecipato il presidente Casini oltre al sottoscritto,

Le forze dell'ordine, è stato detto, non percepiscono straordinari e festivi; hanno una indennità di buoni pasto di 4,33 euro, rispetto ai 7,50 euro degli impiegati civili dello Stato. Mi si deve spiegare per quali ragioni gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze dell'ordine devono avere il 40 per cento in meno di rimborso dei buoni pasto rispetto ai propri colleghi

non soltanto di equità, ma di dignità dei nostri servitori dello Stato cui dobbiamo riconoscenza più di altri perché sorvegliano le città e danno sicurezza a noi stessi e ai nostri familiari.

Voglio farvi sapere che nel 2002-2003 il centro-destra stanziò 760 milioni; nel 2004-2005 stanziò 400 milioni; nel 2006-2007, invece, sono stati previsti soltanto 80 milioni e per il 2008 e 2009 non è stato previsto un euro.

ma non si è potuto prevedere niente per le forze dell'ordine, quasi che siano figli di un Dio minore. Non dobbiamo essere solidali soltanto quando partecipiamo ai funerali, dove ci sono tristi circostanze che ci ricordano l'impegno di queste categorie, ma lo dobbiamo essere sempre, anche in questa occasione.

destinando 250, 300 e 350 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Spero che con queste proposte si possa dare una parte di risposte ad un'emergenza che è di tutti e non solo di questa parte politica.

praticamente parlando anche dei nostri emendamenti presentati all'articolo stesso. Qui mi tocca per un attimo fare il leghista, perché veramente si continua a parlare di problemi probabilmente secondari, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica dello Stato, e si continua invece abilmente a glissare sui problemi veri. Qui parliamo di amministrazione dello Stato, con particolare riferimento ai dipendenti pubblici. Allora, mi piacerebbe capire perché in quest'Aula non si parla mai di quanti sono i dipendenti pubblici, che in un posto normale sarebbe la prima cosa che tutti tirerebbero fuori.

la stima più vicina alla realtà è che superano abbondantemente i 4 milioni e, se si considerano tutti i contratti strani che non vengono calcolati, arriviamo alla cifra iperbolica di quasi 5 milioni di persone.

in Inghilterra ne hanno poco più di 2 milioni, che lo Stato federale degli Stati Uniti, con 300 milioni di abitanti, pare abbia più o meno lo stesso nostro numero di dipendenti pubblici, che

ha pensato bene di raccattare qualche voto in più dispensando posti pubblici a destra e a manca, facendo diventare stabili tutti i contratti che stabili non erano e trasformando lo Stato non più in un luogo dove si amministra il bene pubblico, ma semplicemente in un gigantesco stipendificio, senza nessuna relazione tra il costo del personale e i servizi erogati. Anche qui però - come dicevo all'inizio, mi tocca fare il leghista - si fa sempre

numeri, di problemi dell'amministrazione pubblica, cose di cui perlomeno bisogna essere coscienti, poi ognuno tirerà le conclusioni che vuole - con 5 milioni di abitanti, cioè la metà della Lombardia, ha 26.000 dipendenti, cioè ne ha 12 volte di più con metà della popolazione.

fare la scorta alle mogli dei Ministri quando vanno a fare la spesa al supermercato e la parte restante è imboscata negli uffici, noi la sicurezza sulla strada non la avremo mai comunque. In Italia tra Carabinieri,

Nonostante questo, considerato che qualche mese fa abbiamo parlato dei rifiuti della Campania di Bassolino, non mi pare che con meno dipendenti i Comuni padani siano gestiti peggio dei Comuni che di dipendenti ne hanno il doppio o il triplo. Pertanto, bisognerebbe

di spesa pubblica, il che ci mette fuori dal consesso internazionale per sempre se in qualche modo non risolviamo questo problema. Qualunque persona normale, che lavora nelle aziende private (non quelle che prendono 700.000 euro nello Stato a fare non si capisce bene che cosa), segue una regola semplicissima che in tutte le scuole di amministrazione e di organizzazione aziendale viene insegnata, lo *zero based budget*: quando si organizza non si parte dalla pianta organica esistente per ragionare sulle aggiunte, ma si ragiona sul servizio da dare, su quante persone servono, se quelle che ci sono vanno bene si tengono, se non vanno bene si collocano da un'altra parte, spendendo il minimo indispensabile per dare il servizio richiesto. Voi non state facendo assolutamente nulla di

anche tenuto conto dell'esperienza e che il comparto sicurezza e il comparto delle Forze armate stanno insieme anche quando si tratta di fare i contratti. Quando si tratta di fare audizioni e incontri questo, anche nella mente e nel cuore della gente, è un comparto che sta insieme per i compiti delicati di difesa del nostro Paese.

cioè, allorquando ci saranno i concorsi per le assunzioni, con le nuove risorse che il Governo ha trovato in questo triennio, si tenga conto anche dell'esigenza di trovare

al relatore e al Governo, che sono di parere diverso, per rivedere la loro posizione, perché la norma autorizza al Ministero dell'economia e delle finanze una spesa di ben 4 milioni nel prossimo anno e 9 milioni nel 2009 per ulteriori assunzioni di personale, laddove la legge finanziaria dell'anno scorso, la legge n. 296 del 2006, prevedeva la realizzazione di un ampio piano di soppressione di uffici periferici, che lo stesso Ministero ha anche avviato, al fine di conseguire dei rilevanti risparmi di spesa. La norma che proponiamo

resistere. Lo dico da uomo della Campania, non tanto e non solo perché la mia Provincia di Benevento vedrà eliminati e chiusi gli uffici periferici dell'amministrazione del Ministero dell'economia, ma perché questo accadrà anche ad Agrigento, a Ragusa, a una serie di realtà territoriali.

l'attenzione che è stata sollecitata da diversi colleghi su questi temi, desidero fare una considerazione preliminare, in modo da procedere poi in modo spedito. Il testo dell'articolo 93, come è stato ricordato, al comma 4, riserva risorse rilevanti per le assunzioni

di legge finanziaria, con il quale si è provveduto a stanziare risorse molto rilevanti, oltre che per l'Agenzia delle entrate e quella delle dogane, anche per i Vigili del fuoco e la Forestale, per il contrasto all'immigrazione clandestina, per la Guardia di finanza, per la Polizia penitenziaria e così via. Lo stanziamento di queste risorse con l'articolo 7-*ter* consentirà anche di liberare risorse per poter operare ulteriori assunzioni nei Corpi della Polizia di Stato e dell'Arma dei

che mi sembra utile perché attribuisce al Governo la possibilità, nell'indire concorsi per l'assunzione nei Corpi della polizia e dei Carabinieri, di attingere

esposta dal senatore Tofani che mi sembra meritevole di grande attenzione. Mi riferisco al fatto che estendiamo la normativa relativa al collocamento obbligatorio,

Ringrazio il senatore Tofani per aver avanzato questa proposta che ci consente di introdurre nel nostro ordinamento una norma utile. Esprimo

appoggiare l'emendamento 93.6 del collega Galli, ma facendo una precisazione a nome del Gruppo di Forza Italia. A nostro parere, occorre non confondere tra operai forestali, che sono una cosa, e Corpo forestale dello Stato, che è invece tutt'altra cosa.

corpo sono a Roma, presso il Ministero per le politiche agricole, mentre sarebbe opportuno disporli sul territorio a contrastare fenomeni e reati estremamente pericolosi e, per certi aspetti, nuovi, come i reati ambientali, ma anche le truffe comunitarie.

**Il Senato non approva.** Presidente, l'articolo 93, come altri colleghi hanno ricordato, in particolare il relatore, fissa tra l'altro tetti di spesa per l'adempimento di funzioni di ordine pubblico, di prevenzione e di contrasto alla criminalità. L'emendamento 93.9 punta a contenuti incrementi di risorse su fronti così importanti. Ho ascoltato quello che ha detto il relatore, ma forse aveva presente le finanziarie degli anni dal 2001 al 2006 perché effettivamente, in quel quinquennio, le risorse per la sicurezza sono cresciute complessivamente del 30 per cento. Per quanto riguarda la finanziaria 2008, invito chi si suggestiona nella lettura delle tabelle a consultare, se non crede alle mie parole, la Tabella 8, dedicata al Ministero dell'interno.

tabelle, si arriva alle spese per il SISDE. La tabella utilizza ancora il termine SISDE. Informo chi l'ha redatta che vi è stata qualche novità nel frattempo.

e 36 milioni di euro in meno per le spese riservate dello stesso SISDE. Si dice spesso che, a fronte di fenomeni particolarmente gravi ci vuole l*'**intelligence*. Qui ci vorrebbe non *intelligence*, ma intelligenza per rifiutare una finanziaria che massacra in questo modo la sicurezza. Sono grato al Governo e alla maggioranza che, attraverso il relatore, segnala attenzione verso le questioni di sicurezza degli italiani. La prossima volta non ve ne preoccupate: staremmo sicuramente meglio. Di quale risorse aggiuntive si parla se ci sono 840 milioni di euro in meno per il comparto Viminale?

che sono stati un gentile *cadeau* che la Commissione ha fatto a questo testo di legge finanziaria. Infatti, dobbiamo dire la verità, il Governo in questa materia è stato piuttosto sobrio, la Commissione bilancio si è sbizzarrita nel corso dei lavori e ha arricchito taluni articoli, soprattutto questi che sono articoli clientelari,

flessibili con la pubblica amministrazione che urta in maniera clamorosa con le norme costituzionali, con i princìpi generali del nostro ordinamento, con una miriade di sentenze della Corte costituzionale,

se lo hanno superato, lo hanno superato per le esigenze connesse a quel tipo di contratto; ora si troveranno ad essere dipendenti della pubblica amministrazione in spregio a tutte le regole di buonsenso. Credo che l'unico modo di rimediare a questa

il collega Azzollini, però indubbiamente l'impatto con la norma costituzionale è chiaro ed evidente e molti commentatori hanno espresso gravi perplessità su questo punto, proprio perché hanno ritenuto la norma diseducativa, illegittima e soprattutto diretta contro tanti giovani che vogliono affrontare concorsi seri per accedere alla pubblica amministrazione e che si troveranno scavalcati da persone che non hanno superato alcuna prova selettiva o, se l'hanno superata, l'hanno superata per altri obiettivi e con altre finalità. Io mi vorrei rivolgere, Presidente, ai numerosi padri della patria

dal senatore Pastore sono stati oggetto, da parte della Commissione, della maggioranza e del relatore, di un'attenzione particolare

che l'accesso alla pubblica amministrazione avvenga attraverso concorso, corregge esattamente quegli aspetti critici che indubbiamente il testo approvato in Commissione presentava. Talché si procede ad una stabilizzazione

grazie all'approvazione dell'emendamento D'Amico, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali e delle norme di merito che regolano la materia. quindi, rassicurare i colleghi della maggioranza. Grazie all'approvazione dell'emendamento 93802 (testo 2), così come ce l'ha proposto il relatore e così come esso è stato elaborato dal senatore D'Amico, anche quelle osservazioni critiche che molti non solo in quest'Aula, ma anche fuori da quest'Aula (penso, per esempio, all'intervento autorevole del professor Rossi sulla prima pagina del "Corriere della sera") hanno sollevato sono state tenute in assoluta considerazione

superamento della precarietà, ma in perfetta compatibilità - insisto - con l'esigenza di garantire che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione avvenga secondo procedure selettive che garantiscano della qualità e delle caratteristiche del personale che viene assunto. Quindi, nessuna violazione, soltanto coerenza nel perseguire un disegno di stabilizzazione compatibile con i princìpi generali del nostro ordinamento.

che si nasconde dietro la foglia di fico delle prove selettive. Senatore D'Amico, chi ha esperienza di prove selettive in questo Paese sa benissimo cosa significano.

Lei deve togliere la scheda o deve votare in un altro modo. Deve votare in dissenso dal suo Gruppo. Senatore Novi, lei non può fare così! No, non può parlare perché stiamo votando. Lei ha il dovere di votare in dissenso. Senatore Novi, la richiamo all'ordine per la prima volta. Lei deve togliere la scheda o deve votare in un altro modo. Senatore Schifani, la prego di aiutarmi a gestire il senatore Novi. Senatore Schifani, lei è il Presidente del Gruppo e conosce le regole forse meglio del senatore Novi. Senatore Novi, la richiamo all'ordine...

Senatore Novi, la prego di ascoltare un momento la mia risposta. Abbia la cortesia di ascoltarmi. Lei può sindacare politicamente il comportamento parlamentare di alcuni nostri colleghi.

Per il resto, lei ha fatto delle osservazioni che non posso naturalmente accogliere in questa sede in qualità di Presidente.

Scusate, colleghi. Stiamo svolgendo una discussione procedurale delicata e il senatore Castelli sta esprimendo le sue opinioni.

Credo che questa mia tesi sia assolutamente sostenibile e, se invece ci sono dei senatori della sinistra che distrattamente, per levità o perché non hanno ancora capito dove diavolo stanno sedendo, non agiscono in questo modo, allora si ha diritto - come lo ha il senatore Novi - di richiamare tali questioni.

di astensione, cioè 160 voti, da noi irraggiungibili. Se mi fate la cortesia personale di finirla di urlare, forse ne guadagniamo tutti, soprattutto in termini

La questione riguarda lei e la sua conduzione dell'Assemblea. Abbiamo avuto un voto in meno perché lei ha chiesto al senatore Novi di estrarre la scheda.

Credo che lei abbia abusato del Regolamento. Lei ha richiamato due volte all'ordine il senatore Novi. C'è il rischio che al terzo richiamo lei possa prendere un senatore e cacciarlo dall'Aula. Credo che lei, ripensando a quanto è successo, possa anche ripensare a quella sanzione che - per carità - non ha avuto altro esito. Ma non si può fare ad un senatore la parte che lei ha fatto. Perché vede, signor Presidente, quando noi abbiamo contestato la senatrice Rame per l'atteggiamento che ha avuto, non c'è stato il Presidente dell'Assemblea che l'ha richiamata all'ordine per il suo atteggiamento. Come la senatrice Rame... Chiedo scusa... perdite di tempo, a parte il fatto che sono sgradevoli per la Presidenza e ovviamente per il senatore Storace, che adesso sta intervenendo. Stiamo svolgendo una discussione procedurale: la vogliamo concludere o no, questa discussione? La prego, senatore Storace, prosegua. signor Presidente, noi abbiamo contestato l'atteggiamento della senatrice Rame, l'altra parte del Parlamento dice che ha fatto bene: sono opinioni.

Senatore Nania, cerco di essere attento, abbiamo segnato tutti coloro che intendono intervenire. Senatore D'Onofrio, mi scusi, diamo la parola al senatore Nania.

Si rende conto delle conseguenze assurde che avrebbe la sua interpretazione? Il voto è un fatto personale del senatore Novi, estremamente e soltanto personale. Lei non può assolutamente impedire ad un parlamentare,

che non va tenuto né nei confronti del senatore Novi, né nei confronti della senatrice Rame, né nei confronti di ciascuno di noi che abbiamo tutto il diritto, come si conviene in un normale rapporto democratico, di fare ricorso a tutti gli strumenti che l'opposizione consente

a votare per forza nel modo indicato. È una lesione della facoltà che ciascuno ha di cambiare opinione tra la dichiarazione di voto resa e il voto effettivo che va ad

per ragioni complessive, le regole procedurali talvolta sono interpretate con saggezza dai Presidenti di turno per evitare che si traducano in fatti, per così dire, odiosi,

lo dico perché il voto in dissenso è stato immaginato nel Regolamento del Senato, come immagino in quello della Camera, per garantire politicamente il dissenso di ogni parlamentare rispetto al proprio Gruppo,

ha ritenuto opportuno, in vista del conseguimento di un risultato unitario nello svolgimento dei nostri lavori, concedere ai Gruppi di opposizione, qualunque sia la loro consistenza, un'ora di tempo in più rispetto a ciò che era stato indicato al momento del contingentamento. Da questo punto di vista,

opportuno far prevalere la saggezza rispetto alla rigidità delle regole. In questo modo il Senato ha funzionato e laPresidenza dell'Aula ha consentito di farlo funzionare regolarmente. Se il collega Novi ha votato togliendo la

In questo momento preferisco che l'Assemblea si affidi alla saggezza del Presidente di turno, quale che esso sia, e in questo caso alla sua saggezza, utilizzando il tempo dei senatori di ogni Gruppo mettendolo a carico del proprio Gruppo, al di là delle intenzioni che esprimono.

Presidente, vorrei riportare un po' di serenità e fornire un ulteriore elemento di conoscenza a lei e all'Aula su ciò che è accaduto.

un uso distorto dello strumento di voto in dissenso, dato che questo tutela il dissenso reale e non è uno strumento per guadagnare tempo rispetto alle decisioni dell'Aula condivise sulla distribuzione dei tempi. Avrei compreso di più la sua decisione e la sua fermezza nel richiamare all'ordine il senatore Novi se si fosse determinata un'iniziativa, da parte dell'opposizione, di abusare di questo strumento. In realtà eravamo invece in un momento in cui nessuno

il mio *pressing* dell'ultimo istante e probabilmente la sua sanzione è stata troppo severa rispetto a quello che stava capitando. La ringrazio per l'attenzione.

ho ritenuto di aderire al suo richiamo di invitare il collega Novi ad essere conseguente con la dichiarazione di voto;

proprio per questo fine ho preferito richiamare io il collega Novi (non richiamandolo sotto il profilo disciplinare, ma invitando il collega Novi a sfilare la scheda) scheda) per evitare che in Aula si realizzasse l'attivazione di un provvedimento che non avrei condiviso e che le avrei contestato. Dico questo perché riconosco che è prassi parlamentare dico prassi - che, in presenza di un voto in dissenso, poi quel voto si realizzi conseguentemente in coerenza al dissenso manifestato; ma si tratta di prassi,

non sia una cosa ammissibile. Abbiamo assistito a scene forse mai realizzatesi in quest'Aula di votare contro propri emendamenti. Ci troviamo dinanzi ad un aspetto costituzionale e ad un aspetto di prassi. Costituzionalmente qualunque parlamentare, fino al momento in cui non manifesta la sua volontà con il voto, è libero di cambiare idea rispetto a quella manifestata precedentemente.

al senatore Novi doveva essere consentito di manifestare in ogni caso il suo voto, salvo poi - diritto della Presidenza, da un lato, e diritto del Gruppo, dall'altro - azionare determinate procedure, determinate riflessioni per quanto atteneva all'anomalia del comportamento del collega; ma sono due aspetti diversi due aspetti diversi che attengono a livelli diversi, altrimenti mi dovrei lamentare del fatto che la Presidenza di turno non abbia imposto alla collega Rame di votare il proprio emendamento. o si è coerenti su tutto, Presidente, o non lo si è. Mi auguro che la mia riflessione possa concludere questo dibattito, perché mi assumo la responsabilità di avere invitato il collega Novi a sfilare la scheda, proprio perché ho voluto evitare incidenti d'Aula. Dal momento che alcuni suoi colleghi di maggioranza hanno sostenuto, con dichiarazioni pubbliche, che qui si voleva fare «ammuina» oppure ostruzionismo per impedire il voto della finanziaria, poiché siamo abituati a queste accuse strumentali, mi sono caricato di questa responsabilità, ma solo per far apparire all'intero Paese che, anche dinanzi a comportamenti anomali, non ci stiamo, non abbocchiamo e intendiamo andare avanti nel nostro percorso di grande responsabilità.

poiché stiamo anche abbastanza attenti al dibattito, ci sembrava che anche il collega Morando avesse fatto una dichiarazione sulla falsariga del collega Novi, dichiarando cioè di votare in dissenso dal suo Gruppo. Ciò non è avvenuto e non ci pare che lei abbia usato lo stesso metro di valutazione, non ha chiesto cioè al senatore Morando di sfilare la scheda o di votare in modo conforme alla sua dichiarazione. Volevo solo evidenziare questo aspetto, che magari è sfuggito a chi era un po' più distratto in Aula.

mi meraviglia questa sua osservazione. BUTTIGLIONE *(UDC)*. Lei ha ordinato ad un senatore di votare in un modo piuttosto che in un altro: questo è inammissibile e non può costituire precedente. Lei aveva titolo

onorevoli colleghi, ritengo che esprimere un dissenso dal proprio Gruppo sia una cosa molto seria, non facile e che richiede una partecipazione e un confronto. Credo che giustamente in quest'Aula sia prevista la dichiarazione in dissenso dal proprio Gruppo, proprio per garantire l'autonomia e il rispetto della coscienza e della volontà di ogni singolo senatore.

perché l'articolo 66 del nostro Regolamento dice che «Se un senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale».

La questione è nata sia alla Camera che al Senato perché, ad un certo punto, nei casi di ostruzionismo dell'opposizione, a prescindere dal colore, tutti i colleghi intervenivano ovviamente in dissenso, occupando uno spazio infinito per ogni emendamento. Allora si è stabilito

alcune argomentazioni. A parte qualche forzatura, si capiscono gli espedienti dialettici. Paragonare il voto in dissenso di un collega che ha

ma, nel momento in cui ci sono delle regole supportate anche dalla prassi, il comportamento non può essere diverso da quello che lei ha adottato.

Probabilmente l'estrazione della scheda era il male minore per il collega Novi e quindi mi pare che lei abbia suggerito il male minore, però, oggettivamente, avremmo dovuto lasciare al collega Novi la possibilità di scegliere se votare contro o se astenersi, oltre che se ritirare la scheda. Certo è, però, che lui non poteva votare così come aveva dichiarato il rappresentante del suo Gruppo.

di ciascuno. Accolgo quindi l'invito a questa riflessione. Devo dire francamente che delle osservazioni critiche che sono state fatte circa la posizione assunta dalla Presidenza al momento della votazione dell'emendamento precedente, con riferimento in particolare al voto del senatore Novi, ce n'è una che mi ha particolarmente

addirittura da un atteggiamento quasi intimidatorio nei confronti del collega, di imporre il voto. Non è stato così, non solo perché non è mia intenzione o mio costume imporre niente a nessuno (lo posso assicurare al senatore Buttiglione, anche perché se fosse così sarebbe una delle cose di cui mi vergognerei), ma anche perché la mia iniziativa è stata motivata, a mio modo di vedere, da una questione molto semplice. Collega Boccia, io non ho rispettato una prassi

2, è scritta una cosa molto precisa: tutti i senatori hanno diritto di parlare, anche dopo che c'è stata un'espressione di dichiarazione di voto da parte del Presidente del Gruppo, o comunque di un delegato del Presidente a dare un certo parere su un determinato provvedimento a nome del Gruppo medesimo. In quel momento del dibattito il diritto alla parola, il diritto alla parola, cioè il diritto a prendere la parola su quell'argomento da parte del parlamentare - in questo caso del senatore - è subordinato alla dichiarazione di dissenso. Questo sta scritto nel nostro Regolamento. Io ho ripetutamente chiesto al collega Novi se il suo intervento era in dissenso il collega Novi ha risposto che il suo intervento sarebbe stato un intervento in dissenso. Non mi ha chiesto la parola per un richiamo al Regolamento o sull'ordine dei lavori; mi ha chiesto la parola per intervenire in dissenso dal suo Gruppo. Lo ha dichiarato il collega Novi. Possiamo verificare i resoconti della seduta per constatare questa affermazione. Nel momento in cui siamo andati all'espressione del voto, il collega Novi, contraddicendo ciò che egli aveva detto e non ciò che io avevo imposto, ha votato e insisteva per votare in un altro modo.

posso assicurare i colleghi che lo spirito della Presidenza è stato quello di interpretare la lettera del Regolamento, non una prassi. Dopodiché, senatore Novi, lei avrebbe dovuto chiedermi la parola

della questione della stabilizzazione sugli specifici aspetti di copertura. Già in altre occasioni abbiamo visto quali e quanti elementi ci sono di scopertura in questa finanziaria; questo è un altro di quelli che a me paiono macroscopici. Approfitto della presenza del Ministro per sottoporglielo sommessamente, ma convintamente, tenuto conto che egli, naturalmente, in più sedi - nazionali ed internazionali - presenta questa come una finanziaria di rigore. Chiederò com'è possibile che si continui, dopo l'approvazione di queste ulteriori norme, anche nella versione emendata dal senatore D'Amico, sulla quale dopo si discuterà, a parlare di finanziaria di rigore. Ricordo a tutti, a me stesso primo di ogni altro, che questa procedura per intero è cifrata 20 milioni di euro l'anno.

legislatura, basterebbero a mille persone. Perché? Semplice. Si afferma sempre, quando si parla di stabilizzazione, che siccome

euro. Quindi, la norma è clamorosamente scoperta. Ma, volendo essere buoni con questa maggioranza (considerate le enormi difficoltà che ha a procedere ed a legiferare, l'opposizione tenta di essere buona),

con la stabilizzazione e supponiamo che questo sia di 2.000 euro all'anno, cioè di 150 euro al mese, 130 con la tredicesima. Parliamo di 10.000 precari.

in realtà, con una serie di giri di parole parlate di progressiva stabilizzazione, di norme e di altro, tentando cioè di porre dei paletti di ingresso,

(guardate che è accaduto per altri settori del precariato, penso alle famose borse di studio degli studenti in medicina)? Accadrà che i precari saranno costretti a far causa allo Stato e alle amministrazioni locali per ottenere la stabilizzazione che altri hanno forse nel frattempo avuto - e moltissimi invece no - e a quel punto sarete costretti ad ammettere gli stessi precari in un tempo più lungo, gettandoli nello sconcerto. Cioè, state facendo entrambe le cose: avete certamente devastato il bilancio e non avete soddisfatto le aspirazioni della gente. Così il vostro è stato un disegno perfettamente riuscito:

questione. Quella norma, lo dite testualmente, è prevista per tre anni: 2008, 2009 e 2010; non dite «a decorrere dal», per cui non si capisce com'è possibile

Ritengo invece che, a sua volta, quell'emendamento, attraverso l'inserimento delle questioni relative agli enti locali, può comportare un ulteriore allargamento della platea, con i difetti che ho detto prima. Cosa state combinando con questa norma è cioè del tutto evidente. Vi voglio dire - ed ho terminato - che se le stime fossero di 200.000 precari - sono stime prudenti queste che cito perché altri li fanno ammontare, tra quelli dello Stato e quelli degli enti decentrati, a 400.000, ma io, come al solito tenero verso questa maggioranza che incespica di ora in ora, cifro in appena 200.000 - pensate questa norma cosa costa al bilancio dello Stato. Non mi pare che voi stiate facendo del rigore. È ovviamente chiaro che dovreste avere il coraggio,

andando di questo passo stiate contravvenendo a tutte le vostre dichiarazioni e ad ogni comportamento sano per l'economia della Nazione.

93.801 e sento l'intervento di Azzollini, c'è qualcosa che non funziona: o lui non l'ha letto oppure

il problema dei precari nella pubblica amministrazione, inserisce una norma che, attraverso concorsi, riserva il 50 per cento dei posti

esattamente con 20 milioni. Io ho sentito il senatore Azzollini parlare di questi 20 milioni, riferendosi probabilmente al

io credo che l'emendamento, quanto valutato in Commissione più l'emendamento D'Amico - sul quale si è costruito nelle settimane passate un can can

nella pubblica amministrazione, non si possa più assumere se non attraverso concorsi e personale a tempo indeterminato e prevede di trovare delle norme che si raccordino a quanto previsto dalla finanziaria dell'anno scorso e attraverso le quali si possa procedere ad una stabilizzazione, cioè ad uno smaltimento del problema attraverso regole precise, sempre attraverso concorsi e con riserve di posti di molto inferiori a quelli previsti dall'opposizione, con l'emendamento Azzollini. Addirittura, per quanto riguarda la questione dei Co.co.co.

credo che da parte dell'opposizione ci voglia un po' più di coerenza. Non si possono presentare emendamenti che dicono una cosa e accusare la maggioranza di fare delle «porcherie» - come viene detto - di portare allo sfascio i conti pubblici e lo Stato e poi presentarne altri che vanno esattamente nella direzione opposta,

che l'opposizione voleva risolvere il problema dei precari e la piaga dei precari ma non ha potuto per colpa della maggioranza che non ha approvato il loro emendamento.

il ministro Padoa-Schioppa, che penso non sia venuto qui soltanto per fare un giro ma - immagino - anche per interloquire con il Parlamento,

- si stabilizzano anche tutti gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, Quali sono questi enti in cui c'è veramente un bisogno incredibile di stabilizzazione? La Cassa depositi e prestiti, dove ci sono un sacco di precari, ovviamente tutti iscritti ai sindacati di sinistra, la Zecca dello Stato, l'Istituto poligrafico. Giusto. Dovete regolarizzarli perché servono per attirare i soldi per coprire le spese perché con 20 milioni di euro non so come si faccia. Poi però si vanno a regolarizzare anche quelli dell'ENAC; va bene, se sono 1.000. Vi sto facendo l'elenco di quelli che voi stabilizzate. L'Agenzia spaziale italiana mi starebbe bene, anche lì qualcuno ci sarà.

l'ente autonomo per l'Esposizione universale internazionale di Roma del 1941. Bene, c'è bisogno di stabilizzare anche lì; c'è infatti un bisogno di sicurezza in questo ente fondamentale per il futuro del nostro Paese. Ora vorrei chiederle, signor Ministro, ma chi paga per queste 400.000 persone? Paga la Padania, ma pagheranno tutti. Lei contrae un debito con il futuro che pagheranno i nostri figli. Questo è irresponsabile e mi rivolgo a una parte di questa maggioranza che ha limitato il danno al 2008-2009: ma voi fate salvi i contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Ma quante sono queste persone che promettete di stabilizzare? Ce n'è veramente bisogno? Quanto costano? Signor Ministro, in Europa qualcuno l'ascolterà.

avuto quando ha usato delle espressioni pesantissime e violente nei confronti del generale Speciale, quando ha adoperato espressioni pesanti e violente per giustificare la rimozione del consigliere Petroni dal Consiglio ma lo abbiamo avuto poche volte quando gli abbiamo chiesto di darci chiarimenti sulla politica economica del Governo.

ci eviti per l'ennesima volta i suoi sorrisini irridenti e provocanti nei confronti dell'opposizione. Limiti i suoi sorrisi, faccia il Ministro. Eviti di sbadigliare, di lasciarsi andare ad atteggiamenti quasi ostili a quello che è il ruolo di quest'Aula. Sbadigli di meno,

che meritano tutela, ma che non hanno vinto nessun concorso, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Ministro, si assuma le sue responsabilità e ci spieghi per quale motivo state realizzando questa oscenità.

prego, senatore quest'Aula ha verificato, la settimana scorsa, la totale inadeguatezza del Governo a rispettare le procedure di copertura di tutti i provvedimenti. Tutti voi, tutti noi abbiamo toccato con mano, rispetto al noto emendamento sui *ticket*, che il Governo aveva mentito all'Aula del Senato e che non c'era la copertura.

Perdonate, l'età avanzata giustifica la stanchezza.

ad un costo lordo di 20.000 euro all'anno comprese le imposte e i contributi sociali, si determina un aumento annuo delle spese di personale nella pubblica amministrazione pari pari a 4 miliardi di euro. Se fossero 350.000, tale spesa salirebbe a 7 miliardi di euro.

Se i precari già lavorano, vuol dire che l'attuale costo a bilancio dello Stato è almeno il 50‑60 per cento di quello che avrebbe a regime. E allora lei, onorevole Tecce, ha dichiarato all'Assemblea del Senato che l'articolo 93

perché la copertura data nel provvedimento è pari a 20 milioni di euro. Quindi, la stabilizzazione su base aritmetica basta per 2000 persone, altro che 200.000. voi della sinistra alternativa state stabilizzando 2000 persone e dimenticando gli altri 198.000, dal vostro punto di vista. Concludo, signor Presidente, il Ministro dell'economia, presente in Aula, è persona capace di fare ben di più delle operazioni aritmetiche:

Presidente, avrei voluto prendere la parola

la discussione che si è sviluppata intorno a questi emendamenti evidenzia la politica del Governo. Vede, signor Presidente, sono stati

non vede di buon occhio la libera intrapresa, una finanziaria che nega persino i fondi agli emotrasfusi che hanno dovuto subire danni in forza di trasfusioni dovute a pesanti malattie e che adesso finge di stabilizzare i precari per fare un'operazione di propaganda che purtroppo non trova senso nelle cifre, come hanno evidenziato i colleghi.

ad emendamenti che non costavano una lira, come quello sulla specificità degli uomini in divisa, che non sarebbe costato nulla se non la buona volontà da parte del Governo di indicare - come ha fatto nel Documento di programmazione economico-finanziaria - che questi signori in divisa esistono e che a questi signori chiediamo prezzi importanti. per non volermi soffermare per forza sull'argomento di cui mi occupo in qualità di Presidente della Commissione difesa, prendo la parola, agganciandomi alle dichiarazioni del senatore Baldassarri e degli altri colleghi, per sostenere - come hanno fatto loro - che questa è una finanziaria che beffa il Paese.

«Prodi a gennaio dia le dimissioni, presenti una nuova lista di Governo possibilmente applicando la Costituzione, cioè scegliendo lui tra i partiti e non lottizzando»;

su un emendamento. Sono stati richiamati all'ordine tutti a prezzo e a suon di provvedimenti miliardari. Ebbene, avrei voluto prendere la parola per dire che, pur avendo pur avendo presentato un emendamento *bipartisan* in occasione della scorsa finanziaria e in questa occasione un altro emendamento solitario sul riconoscimento della specificità del lavoro delle forze dell'ordine e delle Forze armate, che rischiano fino all'estremo sacrificio della vita, anche in questa finanziaria un emendamento a costo zero è stato rimandato al mittente; ma gli emendamenti che costano o che devono beffare il Paese, quelli no, non vengono rimandati al mittente. Allora, non resterò un minuto in più, caro Presidente, in quest'Aula e profitto della verità che è emersa dalla discussione su questo emendamento per abbandonare questo consesso.

che, trionfante, si avvia ad approvarla contro il Paese, contro le classi medie, contro la piccola e media impresa, contro le Forze armate e quelle di Polizia. Non resterò un minuto di più e mi auguro che questa provocazione serva anche alla mia coalizione perché, in mancanza di azioni forti, non saremo in grado di spiegare al Paese perché abbiamo consentito a questa maggioranza di approvare una finanziaria da incubo.

Pistorio, lei insieme ad altri colleghi sta chiaramente disturbando il senatore Palma.

pur accedendo fiduciariamente a quanto detto dai colleghi dell'opposizione, di comprendere se ciò sia vero o no, però credo che a volte giunga il momento delle assunzioni di responsabilità, specialmente quando questo momento è raro nell'ambito della discussione e quest'assunzione di responsabilità viene chiesta una sola volta con riferimento ad una norma specifica.

di allontanarsi dall'emiciclo per consentire al senatore Palma di svolgere il suo intervento.

e l'alzarsi in piedi per esporre in termini chiari il suo pensiero, oltre che un atto di rispetto verso il Parlamento, potrebbe suonare anche come un atto di chiarimento nei confronti di tutti i parlamentari. La scelta spetta al Ministro dell'economia,

chiamano in causa il lavoro che è stato fatto in Commissione, molto approfondito su questo punto, oltreché una corretta interpretazione delle norme aggiunte all'articolo 93, mi corre l'obbligo di fare qualche precisazione, partendo dall'affermazione del senatore Azzollini il quale diceva che o si prendono in giro i precari o si sfascia il bilancio dello Stato in rapporto alla copertura recata dalle norme di cui stiamo discutendo. Non dico nulla sul fatto che - come diceva correttamente il senatore Tibaldi senatore Stracquadanio contiene un'estensione notevole delle possibilità di stabilizzare i precari. Le osservazioni sono le seguenti: in primo luogo, i 20 milioni annui che vengono recati nella copertura sono aggiuntivi rispetto al fondo stanziato lo scorso anno, che ancora non viene utilizzato - per quel che ci risulta - se non in minima entità. luogo, il testo della norma attribuisce alle pubbliche amministrazioni non l'obbligo, ma la possibilità di procedere alle stabilizzazioni.

i requisiti, che vengono ridefiniti con queste norme, non viene attribuito - com'è noto - un diritto soggettivo, non vi è la possibilità di pretendere la stabilizzazione; è in facoltà delle pubbliche amministrazioni disporre o meno, sulla base delle regole loro assegnate, la stabilizzazione. Terzo ed ultimo argomento: le Regioni, gli enti locali e gli altri enti sottoposti al Patto di stabilità, com'è noto, devono rispettare le le regole di programmazione nelle assunzioni e devono muoversi e agire sotto il profilo finanziario dentro i saldi finanziari che sono definiti dalla legge finanziaria. Ciò significa che sulla base di queste regole hanno la possibilità di stabilizzare; non lo fanno attingendo al fondo dei 20 milioni, ma attingendo alle risorse di cui dispongono in virtù delle norme del Patto di stabilità. Piuttosto i colleghi dell'opposizione dovrebbero chiedersi e spiegarci motivo negli anni passati, a fronte del reiterato blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e delle regole che sono state poste e che quest'anno vengono rettificate sulla stipula dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, si è determinato un rigonfiamento enorme di precari nelle pubbliche amministrazioni. Questa è una delle tante eredità di cui stiamo cercando con fatica di farci carico.

ci chiediamo però per quale motivo il ministro Padoa-Schioppa, che non ha alcun dovere di scuderia perché non deve votare non essendo membro di questo Parlamento, sia qui e rifiuti di rispondere alle domande legittime che gli vengono rivolte dall'Assemblea, lasciandosi coprire, dal punto di vista professionale, dal senatore Legnini, che noi tutti ringraziamo. Vorremmo sentire dalla viva voce del ministro Padoa-Schioppa

una discussione che fa riferimento, se vogliamo essere precisi, ad altri emendamenti, per non dire all'intero articolo.

criticato la misura disposta dalla Commissione bilancio, che ha modificato significativamente il testo originario proposto dal Governo. Il senatore D'Amico aveva presentato invero due emendamenti, l'uno più radicale (anche se il termine può essere un po' eccessivo), perché proponeva la soppressione delle modifiche introdotte dalla Commissione e il ritorno al testo originario del Governo, il secondo, successivamente modificato nel testo che ora è al nostro esame, con la pretesa - sembrerebbe - di razionalizzare significativamente le disposizioni che sono state varate dalla Commissione. È con sincera amarezza, senatore D'Amico e colleghi senatori, che devo invece constatare e sottolineare con gli argomenti che velocemente esporrò

la situazione. Collega D'Amico, lei ricorda - l'ha detto poca fa il relatore, senatore Legnini - che questa norma deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cioè la legge finanziaria dello scorso anno, che ha innescato questa operazione che qui viene ulteriormente incoraggiata e solo -come abbiamo visto - debolmente rifinanziata dai ridicoli 5 milioni di euro agli ulteriori 20 milioni di euro, a fronte di una spesa

Questo per dare l'idea delle dimensioni. Ma soprattutto mi consentano lei e i colleghi di rilevare in ordine i problemi sollevati. Per la proposta del senatore D'Amico in qualche misura ricostruisce la corretta priorità che dovrebbe essere riconosciuta ai 70.000 vincitori di concorso e ai 100.000 idonei che attendono - come rilevava poco fa il presidente Schifani - una legittima assunzione. La proposta del senatore D'Amico in qualche misura afferma questa priorità? No. La proposta del senatore D'Amico non risolve il problema fondamentale che darà luogo ad un legittimo ricorso di costituzionalità da parte dei molti cittadini che hanno maturato un diritto e che verranno esclusi. il secondo punto, la proposta del senatore D'Amico garantisce effettive procedure concorsuali per coloro che verranno stabilizzati? Assolutamente no, perché la proposta del senatore D'Amico parla di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e, in ogni caso, fatte salve le procedure di stabilizzazione, quelle generose di cui alla legge finanziaria dello scorso anno, che va letta in combinato disposto con questa norma. Le procedure sono opache, cioè conosciute a pochi, e sono ridicole perché consistenti normalmente nella declinazione del nome e del cognome e di ben poco altro, nel momento in cui si realizzava un colloquio per tutti coloro che sono stati presi con rapporti di collaborazione o comunque con rapporti a termine nelle varie modalità ben note. Tutti costoro hanno superato una prova selettiva, ma molto lontana dalla trasparenza nell'annuncio del concorso e soprattutto dalle complesse modalità che giustamente caratterizzano un concorso pubblico comparativo fra più soggetti, fra i molti che sono stati chiamati ad una prova concorsuale per un contratto di lavoro a tempo indeterminato. tempo indeterminato. Quanti hanno deciso, pur avendo appreso di questa prova selettiva, di non parteciparvi, perché non interessati ad un rapporto a termine, hanno poi partecipato al concorso per un rapporto a tempo indeterminato hanno vinto quel concorso, hanno rinunciato alla prova selettiva. Oggi costoro che hanno fatto quella scelta - giusta giusta in teoria - di rivolgersi al concorso pubblico a tempo indeterminato e, ahimè, di vincerlo, sono danneggiati perché al loro posto andranno coloro che hanno superato

l'80 per cento dei precari sta nelle amministrazioni regionali e locali, le quali sono con certezza considerate tra le amministrazioni che possono procedere. Senatore Legnini, quel "possono procedere"

non devo consumare dichiarazioni di voto in questo senso, ma solo chiarire rispetto al mio reingresso in Aula, che non vorrei venisse equivocato. La coalizione della quale il mio movimento - Italiani nel mondo - è parte, in questo momento mi ha chiesto un atto di responsabilità. *(Ilarità tra i banchi della di permanere fuori da quest'Aula quale clamoroso atto di dissenso nei confronti di una pessima finanziaria, ma sono qui a votare con i miei

dall'emendamento 93.802 (testo 2) ha un elevato contenuto tecnico. Proverò ad essere il più semplice possibile partendo dai fatti, che pure dovrebbero in qualche caso prevalere sulle opinioni. Il fatto di partenza è che negli ultimi anni nelle pubbliche amministrazioni si è creato un vastissimo precariato. I numeri riportati ora dal senatore Sacconi, i più pessimistici, parlano di 400.000 unità, mentre un'altra collega, non ricordo quale, ha parlato di 200.000 unità.

perché quel precariato ha due effetti sulla pubblica amministrazione: il primo è che spesso è stato lo strumento attraverso il quale si è sfondata la finanza pubblica, si è accresciuta la spesa pubblica. L'altro effetto, secondo me non meno grave, è che molto spesso è stato uno strumento non solo per politiche clientelari ma per mortificare l'autonomia dei pubblici impiegati, costretti a subire di volta in volta il ricatto del politico di turno che dice di Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).* Credo che noi che stiamo applaudendo dovremmo riflettere in generale sull'autonomia del pubblico impiegato nonché sulla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Ma, certo, il precariato produce questi effetti.

Introduce un principio secondo il quale l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale ovvero previste dalla legge.

Si dice ora che quel principio non è sufficiente. Ce ne vorrebbero di più rigorosi. Non ho visto questi emendamenti per il maggior rigore e non ho visto il rigore nel momento in cui si procedeva all'allargamento del precariato. A me pare - lo ripeto - che questo sia un buon principio. La seconda questione. Viene espressamente escluso che possa accedere alle procedure di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione dei politici. Cosa vuol dire? I Gabinetti dei Ministeri, delle amministrazioni, degli degli assessori regionali, dei sindaci, dei presidenti di Provincia. Non ho nulla contro le persone rispettabilissime che lavorano presso i Gabinetti, ma deve essere chiaro che quelle persone sono chiamate in funzione di un rapporto fiduciario con il politico di turno ed il loro incarico presso la pubblica amministrazione finisce in quel momento e non si deve neanche immaginare che in quel periodo stanno cercando di trovare l'impiego stabile nella pubblica amministrazione.

Confesso che sono contrario a tutte le riserve. Quindi la mia proposta è di cancellare quella riserva. A me pare ragionevole quanto viene qui previsto che le amministrazioni possano, nel momento in cui bandiscano concorsi, riconoscere l'esperienza ed il lavoro svolto dalle persone. Normalmente vi è in tutti i bandi di concorso. Si potrebbe fare anche se non fosse scritto. Mi sembra giusto scriverlo ma stiamo parlando di questo e non mi sembra un grandissimo privilegio. E vengo alla questione relativa - e chiudo davvero - agli oneri finanziari. Ho sentito contemporaneamente due contestazioni alla norma: la prima è che costa tantissimo e regolarizzerà centinaia di migliaia di persone. La seconda contestazione: non si regolarizzerà nulla. Ora, è impossibile che le due cose valgano insieme, solo una delle due può essere vera. Rispetto a ciò,

cifra determina il limite delle risorse disponibili. Riguardo alle amministrazioni locali, come tutti sappiamo, per motivi vari, siamo costretti addirittura ad imbracarle (francamente,

Non lo dico ironicamente, ma per il contributo di chiarezza che egli ha dato al dibattito ed al confronto su un tema di grande rilievo, che non è complicato dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista sociale ma dal punto di vista sociale e delle aspettative di centinaia di migliaia di persone. Lo dico perché il senatore D'Amico ha fatto uno sforzo, con il suo emendamento, di estetica procedurale e, con il suo intervento, di etica procedurale, ma non ha affrontato il problema vero. Senatore D'Amico, il problema vero è che dopo il suo intervento abbiamo tutti capito che, anche grazie al suo emendamento, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che stabilizza non i precari, ma le aspettative.

perché l'operazione che state compiendo è questa. Se infatti si parte dal numero dei precari, si individua l'assenza di copertura; se si parte dal limite di copertura, si capisce la dimensione numericamente limitata dell'intervento. Il senatore D'Amico ha detto che abbiamo 20 milioni aggiuntivi...

più 5), conoscendo lo stato della finanza locale, stiamo determinando un'operazione che riguarda qualche centinaio di precari, tutt'al più qualche migliaio. Ecco perché parlo di stabilizzazione delle aspettative, perché voi in questo modo state costruendo un bacino. A parte le questioni di ordine tecnico‑giuridico poste dal collega Sacconi, voi state creando un bacino, state sindacalizzando il bacino dei precari, che poi dovrà fare un'enorme pressione per tentare di risolvere il problema di tutti. Vi ricordo che tutto questo è nella storia del clientelismo di massa del centro-sinistra. *(Applausi dai Senatrice Calipari e senatrice Mongiello, statemi a sentire e se avete argomentazioni contestatemi, perché io intercetto la vostra protesta, ma non

e avete determinato enti locali privi di qualità, privi di capacità, privi della possibilità di rispondere alla sfida dello sviluppo,

voi state creando una mina sociale, una bomba ad orologeria, che interverrà in maniera devastante a prescindere dai conti e dalla tecnica. *(Applausi

mi rivolgo in particolare al senatore D'Amico, perché vi è una modifica sostanziale tra l'emendamento originariamente proposto da lui e il cosiddetto testo 2. Lo dico perché si tratta di questioni molto importanti. D'Amico ha detto ripetutamente, e la stampa ha riportato questa sua opinione, che ritiene che la Costituzione preveda il concorso come legittimazione necessaria per accedere ai pubblici uffici.

è casuale che lo sia): «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Lo dico ai colleghi presenti che immagino sappiano che differenza c'è tra il concorso e le procedure selettive di natura concorsuale, che sono acqua fresca o sono altra cosa.

Il Gruppo dell'UDC non ritiene che il precariato di per sé sia una cosa rispetto alla quale essere indifferenti. Il senatore Baccini ha dimostrato come si può contemporaneamente essere severi per il merito e attenti alle questioni della giustizia sociale. Questo è l'equilibrio che noi dovevamo trovare

che la stabilizzazione è subordinata alle procedure selettive di natura concorsuale, fermo restando il principio costituzionale del concorso. Quel principio costituzionale non esiste più. dice che si accede alle pubbliche amministrazioni con procedure selettive. Tutti sappiamo che le procedure selettive possono essere cose diverse dai concorsi in senso stretto, perché l'esperienza concreta ha dimostrato che è così. Allora la questione molto semplicemente è questa: D'Amico concorre alla presa in giro di una stabilizzazione che non avviene, e da questo punto di vista diventa corresponsabile dell'inganno che si perpetra a danno di queste persone persone che lavorano nella pubblica amministrazione, oltre che corresponsabile di una norma manifesto alla quale non corrisponde alcun contenuto reale. Ed è un problema serio che è più interessato al voto della finanziaria e all'inganno politico che non alla garanzia della Costituzione. Si tratta di una questione molto delicata, cari colleghi, molto delicata

quindi, a rendere applicabile a costoro questa sua nuova disciplina legislativa? Delle due l'una: o non si applica a queste persone la procedura di stabilizzazione

siamo contrari ad un emendamento farsa che si illude di cambiare la Costituzione che rimane in vigore. Da questo punto di vista, voglio sia chiaro e che in questo Senato qualcuno ricordi che l'emendamento D'Amico originariamente rispettava la Costituzione, ma oggi non la rispetta più. Per questo voteremo contro